Il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno G1 e favorevole sull'ordine del giorno G2, condizionato a modifiche che sono state accettate dai proponenti.

Italia Viva-PSI sull'ordine del giorno G2 (testo 2), firmato da tutte le forze politiche. Di questi tempi, quando si raggiunge un accordo tra tutte le forze politiche in materia di salute è sempre e solo una buona notizia. Ringrazio in particolare i presentatori e le presentatrici delle mozioni per il lavoro di mediazione tra le forze politiche, in particolare la senatrice Castellone e le colleghe e i colleghi della Commissione sanità che si sono impegnati per questo ordine del giorno. Parliamo di cure domiciliari e con l'ordine del giorno chiediamo al Governo di aggiornare, tramite l'Istituto superiore di sanità, Agenas e AIFA, i protocolli di cura - o sarebbe meglio chiamarle strategie di cura - per medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di tutte le esperienze. In sostanza, quello che chiediamo è di superare il concetto di vigile attesa per i pazienti Covid all'inizio della malattia. Dopo un anno di esperienza è opportuno dare ai medici lo spazio su una gamma di possibilità di utilizzo di farmaci, antinfiammatori o altri, naturalmente sempre nell'ambito di studi scientifici, come ci ha illustrato ieri il sottosegretario Sileri in riferimento alla circolare di novembre. E lo facciamo soprattutto per i pazienti più fragili, gli anziani e quelli affetti da patologie. Il concetto di base è la presa in carico precoce delle persone che si ammalano. In Italia, purtroppo, abbiamo registrato e registriamo ancora troppi morti; una delle cause probabilmente è l'eccessiva ospedalizzazione e, quindi, è molto importante - direi fondamentale - la presa in carico precoce dei pazienti. Mentre l'Italia è impegnata nell'accelerazione della campagna vaccinale, con un piano più ordinato che parte dalle priorità per età e unico su tutto il livello nazionale, ci sono, purtroppo, ancora tante persone, tante famiglie che soffrono per la malattia da Covid-19. Registriamo e intercettiamo anche noi come parlamentari il grido di dolore di quelle famiglie, delle persone che lamentano la solitudine, l'isolamento - il tema più grave di questa malattia è la costrizione all'isolamento - ed è inutile nasconderci che lo registriamo anche in molte lamentele della cittadinanza rispetto all'intervento o meno dei medici di famiglia. famiglia. Per contro, tantissimi sono i medici di famiglia che dal basso - lo ricordava ieri il senatore Romeo - in questo anno hanno costruito anche gruppi spontanei di scambio di esperienze, di di conforto reciproco. Diciamo sempre che i medici sono eroi, ma anche loro hanno bisogno di conforto reciproco, di scambio di esperienze, di buone pratiche dal basso,

di modo che con questo strumento aiutiamo i medici a capire che cosa sta succedendo al paziente. Dovremmo dare le indicazioni di non sospendere ad esempio - per i malati cronici anche in caso di malattia da Covid-19. Dovremmo dare un supporto sociale: non tutti hanno la possibilità di avere abitazioni grandi; non tutti hanno la possibilità di essere accuditi dai familiari.

molto importante. Ma, per stare vicino davvero ai medici, agli infermieri e a tutto il personale socio-sanitario che va nelle case dei pazienti e aiuta a curare i malati, dobbiamo sempre tenere insieme umanità e tecnologia, perché il rapporto umano tra il medico e il paziente è quello più più importante, anche per questa bruttissima malattia. Dobbiamo evitare il deserto che c'è tra la medicina generale e l'ospedale e lavorare per questo. La nostra Commissione è impegnata sul tema della medicina di territorio. Il PNRR del Governo indica alcune soluzioni per avere un presidio territoriale e garantire una continuità assistenziale tra la casa, l'ospedale e viceversa. È l'obiettivo per cui dobbiamo impegnarci come classe politica di questo tempo. Faccio un appello al Governo: a giugno 2020 avevamo già approvato una mozione molto importante sui tamponi, votata da tutte le forze politiche. Probabilmente, se l'avessimo messa in pratica, avremmo evitato di far saltare la la sorveglianza attiva sui territori, anche qui con differenze regionali enormi. Abbiamo imparato - come mi pare abbia detto ieri la senatrice Pirro - alcuni termini che prima erano solo per gli addetti ai lavori, come «tamponi molecolari» o «tamponi In quella mozione già davamo delle indicazioni molto forti e ora lamentiamo il fatto che non sia stata ascoltata. Mi rivolgo allora al sottosegretario Sileri e al Governo: facciamo in fretta ad aggiornare queste cure domiciliari, cerchiamo di avere una sinergia positiva tra Governo e Parlamento su questo tema e diamo seguito subito alla mozione che sarà che sarà votata, appunto, da tutte le forze politiche, perché dobbiamo stare vicino alle persone che soffrono e soprattutto a chi li cura. Se curiamo chi cura, usciremo più facilmente da questa epidemia.

mattina sfugge ai più, in questa modalità un po' intima e un po' distratta dei lavori del Senato, la paradossalità

nel fatto che il Senato della Repubblica raccomanda, sollecita e imprime una spinta al Governo perché faccia direi - quasi il minimo indispensabile del suo dovere, e cioè l'aggiornamento dei protocolli di cura del Covid-19. Stiamo parlando di qualcosa che che rientra nell'ordinaria amministrazione, la gestione di un condominio, del grande condominio di questo Paese, impegnato in un'emergenza che si chiama emergenza da Covid-19, uno strumento indispensabile, quale appunto un protocollo da assegnare alle Regioni e, attraverso le Regioni, a tutto il personale sanitario impegnato nel trattamento della domiciliarità, Noi abbiamo a disposizione oggi un documento del 30 novembre scorso; oggi è l'8 aprile. Nel frattempo sono successe tante cose, anche nelle caratteristiche del virus che circola in modo differente rispetto a prima del 30 novembre. Sono intervenute le varianti, sono intervenuti nuovi farmaci e tutto questo all'insaputa

Dal 30 novembre ad oggi serve il Senato della Repubblica per suonare il campanello e dire «sveglia»: questa è una paradossalità gigantesca, colleghi.

l'attività del Governo Conte, prima, e del Governo Draghi, oggi, in sostanziale continuità. Oggi il Senato della Repubblica si trova a dover dire al Ministro della salute e a tutto l'apparato che lo circonda

una seconda paradossalità e mi dispiace in questo caso dover appuntare un'eccezione rivolta al collega Sileri, che ha letto una relazione evidentemente preparata per lui da qualcun altro.

che fa politica o dovrebbe fare politica. Anche in questo caso ho ascoltato allibito la relazione del rappresentante del Governo e ancora una volta non posso non osservare che siamo totalmente fuori strada. È qui che ci spieghiamo, in modo assolutamente drammatico, perché il Paese le ha sbagliate tutte fino a oggi. Abbiamo il *record* dei decessi

registrato il peggior abbattimento di PIL di tutta Europa e quindi i due provvedimenti, che dovrebbero operare come vasi comunicanti, ovvero le restrizioni per evitare l'aggravamento della pandemia, sono tutti e due al *top*, al massimo

Stiamo fallendo nell'ultima spiaggia, che è quella della campagna vaccinale. Siamo ancora alle prese con la mancanza di vaccini. Anche il decreto Covid tratta

ma un sussulto di dignità, e non mi viene un'altra parola; un sussulto di dignità nel pretendere che questo Governo faccia fino in fondo il proprio dovere, a cominciare dal Ministro della salute che deve affrontare questa pandemia.

e gli dice di aggiornare quella circolare, quel protocollo del 30 novembre scorso, che peraltro

spero che nei prossimi giorni accada più o meno la stessa cosa in tanti altri ambiti: certificata, constatata la limitatezza della capacità di contrasto dell'epidemia, il Senato, per quanto ci riguarda - e la Commissione, per quanto mi riguarda - possa sostituirsi altre volte virtuosamente per integrare le manchevolezze, i ritardi, le lacune

non avendo protocolli a disposizione, hanno cominciato a mettere in pratica approcci su malattie similari esistenti prima del Covid, ovviamente senza avere protocolli terapeutici né dati di fatto e certezze.

Successivamente la comunità scientifica, che non è rimasta inerme, ha cominciato a valutare se almeno per i casi meno gravi fosse possibile anche procedere con una gestione a domicilio, appunto con le cure domiciliari di cui oggi stiamo trattando.

tutto quello che vogliamo, il nostro Sistema sanitario in questa pandemia ha fatto emergere delle criticità che ancora adesso ci sono: il fatto di avere 21 sistemi sanitari diversi che confluiscono in un unico sistema unitario di indicazioni, attraverso anche delle linee-guida omogenee, è molto complicato.

della territorialità non si può non tenere in considerazione. I servizi sanitari sul territorio, quindi, saranno la sfida maggiore per l'applicabilità di queste linee guida nazionali

vista la necessità di armonizzare e sistematizzare tutte le azioni in campo, compreso l'accompagnamento socio-sanitario e il sostegno familiare per fare in modo che nessuno sia lasciato solo, soprattutto le persone fragili, perché ovviamente è quella la categoria che abbiamo sempre in mente di dover sostenere.

sotto controllo. Tutti noi vogliamo che i nostri cittadini, dal Nord al Sud della nostra Nazione, siano curati con le stesse e le migliori le migliori terapie perché possano uscire da questa pandemia, ma sappiamo anche molto bene che è difficile avere omogeneità su tutto il nostro territorio.

diventerà difficile mantenere lo *standard* di 500.000 dosi al giorno per il nostro territorio ed uscire dalla pandemia in brevissimo tempo.

Ieri il sottosegretario Sileri ci ha spiegato, secondo me in modo del tutto apprezzabile, l'attenzione con cui si sta affrontando la questione.

è saltata nel corso degli anni. Se qualcuno volesse guardare con attenzione a cosa è successo negli ultimi anni nella rete territoriale delle diverse Regioni

state messe in discussione la struttura e l'organizzazione territoriali per la presa in carico dei pazienti. Questa questione è rilevantissima. Rilancio una proposta che ho già avanzato in quest'Assemblea e che ora, grazie all'iniziativa di alcune senatrici,

valutando le esperienze sul campo non per dare voti o fare classifiche, ma per capire cosa dobbiamo fare realmente per il *recovery* e come utilizzare al meglio le risorse a disposizione, nonché quale impianto definire, anche dal punto di vista organizzativo, affinché

una crisi economica enorme con oltre 900.000 posti di lavoro persi e la caduta del PIL

ma l'interrogativo che ci dobbiamo porre è: qual è il nostro ruolo? È del tutto comprensibile la tensione presente tra i nostri cittadini,

sia assolutamente pericolosa, soprattutto se chi lo fa ha responsabilità di primo piano a livello istituzionale e sta nella maggioranza di Governo. È molto grave.

si scarichi sul Ministro della salute la responsabilità di questa situazione: è una cosa inaccettabile.

le scelte che si fanno non sono del ministro Speranza, ma sono del Governo, della maggioranza, della Repubblica. Attenzione, perché su questo terreno non vorrei che arrivassero fra un po' di tempo delle lacrime di coccodrillo.

la responsabilità gravissima di fare un danno non a una parte politica, ma all'Italia, al nostro Paese. Vorrei che rifletteste su un punto: stiamo discutendo su aprire o chiudere. La cosa più seria - lo dico personalmente - attendere che i casi comincino a decrescere effettivamente in relazione anche all'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e negli ospedali. Occorre ricostruire il tracciamento, perché in questi mesi - lo sapete tutti

in modo controllato e sicuro. Se avete dei dubbi, guardate quello che sta succedendo in Francia e in Germania.

ultimo punto. Vi propongo di assumere un'iniziativa chiara: l'unico modo per affrontare l'emergenza vaccini è in primo luogo quello di sospendere i brevetti.

che impegna tutto il Parlamento e che quindi speriamo abbia forza presso il Governo per ottenere l'adempimento degli impegni indicati nella nostra mozione, tocca veramente il cuore del problema. Il cuore del problema oggi è che abbiamo scoperto di avere in Italia da un lato una sanità ospedaliera ad altissima evoluzione, anche sotto il profilo tecnologico,

stenta molto oggi a recarsi a casa del paziente e a prendersi cura di lui, anche semplicemente guardandolo in faccia. Molto spesso questa relazione matura e si esaurisce nell'arco di una telefonata;

Cosa voglio dire con questo oggi? Noi dobbiamo ripensare la medicina territoriale, perlomeno sotto tre profili. Il primo profilo fondamentale è quello della competenza del medico di medicina generale. Abbiamo bisogno di restituire al medico di medicina generale una competenza clinica ben più sofisticata di quella che molto spesso assorbe attraverso la tradizionale scuola di medicina. Abbiamo bisogno di sapere oggi (cosa che abbiamo toccato con mano) quanto sa il medico di medicina generale dei quadri come per esempio quello della polmonite interstiziale bilaterale, che ha caratterizzato tutta l'evoluzione della pandemia come elemento di gravità; cosa sa il medico di medicina generale in un contesto formativo che sgancia l'esperienza clinica dall'esperienza più strettamente territoriale? Egli non è esposto alla relazione formativa importante della struttura ospedaliera ad ampio spettro, come quella che dovrebbe garantire la sua formazione sotto il profilo clinico. Abbiamo bisogno di rivedere questa formazione. Sarà inutile spendere tempo ed energie a valorizzare la competenza del medico di medicina territoriale, se non gli garantiamo tutti gli strumenti necessari a raggiungere quella formazione che oggi, considerato il livello sofisticato in cui si muovono le nostre diagnosi differenziali, egli deve riuscire a ottenere. luogo abbiamo bisogno che la medicina territoriale si avvalga veramente di strumenti tecnologici di ultima generazione. generazione. Non possiamo utilizzare strumenti obsoleti e non possiamo sottovalutare la sua formazione sotto il profilo della digitalizzazione.

Oggi una tecnologia sofisticata va trasferita al letto del paziente o comunque a casa del paziente, nel suo domicilio. È lì che dobbiamo portare la tecnologia. Tutti noi siamo abituati a ricevere informazioni e dati sul sul cellulare che abbiamo in tasca, che vibra continuamente mantenendoci, volenti o nolenti, collegati a un filo diretto. Noi abbiamo bisogno che ogni paziente sia, in qualche modo, il centro di una digitalizzazione differita, secondo il vecchio modello *hub per cui si ha una centrale dove si concentrano le competenze di un certo tipo e una distribuzione capillare in tempo reale, cosa che oggi non c'è. Poi, abbiamo bisogno di un terzo elemento fondamentale che è, paradossalmente, l'altra faccia di questa digitalizzazione sofisticata, spinta capillare e diffusiva, che è la qualità della relazione interpersonale. Abbiamo sentito e sappiamo tutti che, per i motivi più vari, molto spesso quella che è venuta meno in questo periodo di pandemia è stata la relazione. I pazienti si sono sentiti soli: si sono sentiti soli perché, in qualche modo, li abbiamo isolati e si sono sentiti soli perché, in qualche modo, si sono isolati. C'è il paziente che si è isolato, all'inizio, per una forma di paura del contagio. Poi, però, questa paura si è trasformata in un'altra cosa, paura di andare in ospedale, cioè la paura di uscire di casa e di non vedere più le persone care. Ci siamo trovati in un contesto rarefatto, in cui il paziente era veramente in una terra di mezzo che non era marcata né dalla medicina

socio-sanitaria. Sono venute meno le istanze che il territorio deve garantire in termini di qualità, di accoglienza e di presa in carico.

molto interessante sulla figura dell'infermiere domiciliare, dell'infermiere familiare. Non è una parte accessoria rispetto a questo progetto, perché anche il medico di medicina generale che lavora sul territorio non può farlo da solo, ma ha bisogno di lavorare con altri, perché ha bisogno di intercettare i bisogni del paziente a 360 gradi e, una volta che li ha intercettati, ovviamente ha bisogno di soddisfarli. Noi oggi sappiamo che il medico guarda in faccia il suo paziente secondo uno stile di formazione clinica, accademica, sociale, organizzativa e tecnologica. Ho detto accademica perché abbiamo bisogno anche di riportare la riflessione scientifica nel lavoro del medico di medicina generale. Se la medicina generale non produce

ma se non faccio senza non potrò prendere decisioni adeguate. Quindi, dobbiamo restituire una dignità molto profonda alla persona, al lavoro e al modello dell'assistenza domiciliare. Dobbiamo investire tecnologicamente e coraggiosamente.

Dobbiamo ripensarla con una *vision* diversa. Non è una medicina di serie B. È una medicina che deve essere di serie A e, per di più, stellata,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la storia ci insegna che in passato l'umanità ha conosciuto molte epidemie e pandemie, ma a gennaio dello scorso anno mai ci saremmo immaginati di viverne una con i drammi e le conseguenze che oggi ben conosciamo. Questo virus, inizialmente sconosciuto, ci ha ricordato la nostra fragilità, mettendo in evidenza la necessità di ripensare a un nuovo modello di sanità. È evidente anche il limite delle politiche basate solo sull'austerità che hanno imposto negli anni passati tagli orizzontali in settori fondamentali come la salute pubblica, e la mancanza di programmazione nelle specializzazioni mediche. Non serve che ricordi i momenti più bui e dolorosi che sono impressi in ciascuno di noi, le tragedie e i drammi che si sono consumati e che ancora oggi si vivono nelle case degli italiani, gli occhi smarriti dei nostri nonni, dei nostri genitori e il senso di impotenza di tanti operatori e medici. Per fortuna, le persone che dedicano la propria vita alla scienza hanno fatto passi da gigante e, unitamente all'arrivo dei vaccini, si è progressivamente adeguata e migliorata la presa in carico dei pazienti. Le conoscenze maturate in quest'anno, grazie alla comunità scientifica e ai medici che hanno anche sacrificato la propria vita, hanno portato a capire che è possibile curare i pazienti al proprio domicilio. La rete territoriale ha avuto e ha un ruolo cruciale con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri che, assieme alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), svolgono un ruolo fondamentale all'interno del tessuto sociale e sanitario, curando i soggetti a domicilio ed evitando l'ospedalizzazione. Ciò che si è compreso è che il Covid-19 continuerà a circolare e, se non si raggiungerà presto l'immunità di gregge, le varianti si moltiplicheranno inevitabilmente. Probabilmente dovremo imparare a convivere con questa situazione ancora per diverso tempo, ma proprio per tale motivo è necessario imparare a gestire la situazione per tornare quanto prima a una vita il più possibile normale, fatta di gesti quotidiani, di lavoro, di relazioni e di rapporti sociali. Di fronte alla consapevolezza collettiva di voler tornare a vivere, vi è la necessità di riformare la medicina territoriale, prevedendo una vera integrazione tra la rete ospedaliera e il territorio al fine di mantenere il più possibile il paziente a domicilio, attraverso un'assistenza altamente avanzata secondo principi di appropriatezza e innovazione. Il Parlamento in questo deve essere protagonista. Ricordo che in 12a Commissione stiamo trattando il futuro e la riorganizzazione della medicina territoriale, che avrà degli indirizzi precisi. Ora è quanto mai necessario e urgente aggiornare i protocolli delle cure domiciliari ormai datate alla luce dell'esperienza sul campo, superando il concetto di vigile attesa e dando la possibilità agli utenti di vedere prescritti i farmaci ritenuti più opportuni, tenuto finalmente conto del singolo caso.

complete e aggiornate alle evidenze scientifiche, cliniche ed esperienziali dei professionisti impiegati direttamente sul campo. Il quadro della situazione è drammatico. Il tribunale del malato conta milioni di visite specialistiche sospese; migliaia di ricoveri non sono stati effettuati; quasi 500.000 interventi sono stati rimandati, mentre oltre 2 milioni di *screening* oncologici sono stati posticipati. Vi è l'urgente necessità di tornare a riavviare la macchina della sanità per far fronte alle altre patologie, che nel frattempo non si fermano, anzi. Per fare questo c'è bisogno di normalizzare il più possibile e velocemente gli ospedali, alleggerendo le terapie intensive e gestendo i pazienti Covid a casa. Questo significa visite domiciliari, rete territoriale efficace, potenziamento della rete diagnostica, rimodulazione del servizio di continuità assistenziale per creare, con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, un vero servizio di continuità assistenziale e di prossimità. Serve la sistematizzazione delle aggregazioni funzionali, sia mediche che pediatriche, anche in microteam, al fine di disporre di adeguato personale amministrativo, infermieristico e ostetrico. Vanno valorizzati i nostri bravi professionisti: i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, protocolli e linee guida che devono tener conto del contributo di chi tutti i giorni cura a domicilio pazienti colpiti dal Covid. che con sobrietà esercitano la loro professione, salvando le vite delle persone e ai quali deve andare il nostro sostegno e il convinto e unanime ringraziamento. oggi intervenire per il mio Gruppo in dichiarazione di voto. Mi sia consentito, nell'anticipare il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, ringraziare tutti i colleghi del mio partito perché tutti, nessuno escluso e ciascuno per la propria parte, sono stati di stimolo nella stesura della mozione sulle cure primarie. Un plauso va al nostro capogruppo Massimiliano Romeo, primo firmatario della mozione sulle cure domiciliari, oggi ricondotta all'ordine del giorno che vede il Senato intero parlare ad una sola voce. al collega Bagnai, che insieme all'assessore Coletto, referente per il nostro partito nell'ambito della sanità, ha presentato gli indirizzi operativi per la gestione dei pazienti Covid-19 in ambito domiciliare. Un grazie va poi alla disponibilità del sottosegretario Sileri, per aver ricevuto l'avvocato Grimaldi, il professor Cavanna e il dottor Stramezzi del Comitato cure domiciliari Covid, professionisti che, come molti altri medici, curano i pazienti a casa. va infine a tutte le colleghe e ai colleghi della 12a Commissione, nessuno escluso, per la disponibilità e la collaborazione. Oggi, come spesso capita quando parliamo di salute, ci ritroviamo tutti uniti. Chiediamo che da domani anche gli enti preposti siano altrettanto celeri e univoci *(Applausi)* nell'aggiornare le linee e i protocolli, così da avere un sistema all'altezza delle aspettative e degli interessi della Nazione. Signor Presidente, sottosegretario Sileri, colleghi, un anno fa ricevevo il messaggio di una delle mie più care amiche, una mia collega del CNR di Napoli. Nel messaggio c'era scritto: «Io non sto bene, ho febbre da una settimana. Appena puoi, chiamami». La richiamai quasi subito e, da come parlava, capii che aveva difficoltà a respirare, affannava. Mi raccontò che aveva febbre da una settimana, che non rispondeva alla Tachipirina e che il medico di medicina generale non aveva potuto visitarla: eravamo a metà marzo, all'inizio del primo *lockdown*.

E così il 118 si recò a casa di Annamaria - questo è il nome della mia amica - misurò la saturazione, trovò che era molto bassa e la ricoverò in ospedale. in ospedale. Qui venne effettuato un primo tampone, ma dopo tre giorni non c'era ancora il risultato, quindi venne effettuato un secondo tampone che diede, purtroppo, esito positivo. Eravamo ormai a tredici giorni dall'inizio dei sintomi. Annamaria allora mi inviò un messaggio vocale - che ancora conservo, come tutti i messaggi di quei giorni - in cui mi diceva: «Sono positiva al Covid, mi stanno trasferendo, non mi abbandonare». Fu trasferita all'ospedale che a Napoli si occupa di curare le malattie infettive e lì finalmente partì la terapia specifica, una terapia antivirale: ma ormai erano passate quasi due settimane dal primo sintomo, quindi quella terapia antivirale ebbe, purtroppo, poco effetto. Fu sottoposta prima alla ventilazione meccanica col casco e poi all'intubazione, e quindi trasferita in un reparto di terapia intensiva dove ha lottato per due settimane. Anche in quelle due settimane ricordo di aver parlato tutti i giorni con i medici di quel reparto: veri e propri angeli che assistono i pazienti con dedizione assoluta.

protocollo poter utilizzare. Ricordo che cercavo di reperire tutti gli studi pubblicati in qualsiasi angolo del mondo per cercare qualcosa da fare, anche di intentato. Non riuscimmo a salvarla e così, il 4 aprile 2020, se n'è andata. Da quel momento ho la certezza che contro il Covid bisogna intervenire precocemente se non c'è risposta alla terapia sintomatica. Con Annamaria eravamo arrivati troppo tardi. In realtà, qualche mese dopo anche il Ministero della salute, in una circolare del novembre 2020, evidenziava come la latenza tra l'inizio dei sintomi, la valutazione clinica e l'inizio della terapia potesse influire sul decorso della malattia. In medicina, quando non c'è la cura per una malattia, il farmaco più potente è sempre il medico: il medico che, con le sue nozioni scientifiche, la conoscenza che ha dei propri pazienti, ma anche con il buon senso, può sempre fare la differenza tra la vita e la morte. A questo riguardo mi viene in mente una frase che mia madre mi ripeteva spesso quando ho scelto di fare il medico; una frase che lei da bambina leggeva nello studio del podestà, che all'epoca era anche il medico del Paese. Ebbene, la frase diceva il medico è colui che cerca, con scienza e coscienza, di portare sollievo a chi soffre. Dobbiamo quindi dare ai nostri medici tutti i mezzi e gli strumenti per assolvere a questo nobile compito. Presidente, mi lasci dire che sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto quest'anno come Parlamento e come Commissione sanità; ringrazio in particolare la nostra presidente, Parente, il sottosegretario Sileri, il ministro Speranza per la loro dedizione e il loro impegno continuo. Grazie al lavoro fatto quest'anno, nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è prevista una vera e propria riforma della sanità che parte dal territorio; quel territorio che è stato l'anello debole nella gestione di questa pandemia, quel territorio che finalmente vedrà strutturate quelle reti di cure primarie e intermedie che finora costituiscano una realtà solo in alcune Regioni. Anche grazie al nostro lavoro parlamentare, finalmente in Italia si utilizzano gli anticorpi monoclonali che sono un'arma importantissima per evitare l'aggravamento della malattia.

si utilizzano i test antigenici rapidi, che ci permettono di diagnosticare ed isolare in maniera precoce tutti i casi positivi e quindi ridurre i contagi. Oggi questo Parlamento dà l'ennesima prova di essere al servizio dei cittadini. Voglio ringraziare, per il grande lavoro svolto in questi giorni, in particolare il collega Romeo, firmatario dell'altra mozione, e lasciatemi ringraziare anche il senatore Zaffini, il collega di opposizione che è con noi in Commissione. Tutti insieme abbiamo lavorato a un testo che chiede quattro cose fondamentali: definire ed aggiornare protocolli e linee guida di cure domiciliari, che siano unitari su tutto il territorio nazionale; coinvolgere tutti gli attori del territorio, quindi non solo i medici di medicina generale e i dipartimenti di prevenzione delle ASL, ma anche gli infermieri di famiglia e tutte le figure professionali; fornire agli operatori sanitari gli strumenti adatti per poter monitorare a domicilio i pazienti, quindi gli strumenti di telemedicina; infine, istituire presso il Ministero della salute un tavolo di monitoraggio di tutti i protocolli che si stanno utilizzando, perché sono moltissimi gli studi clinici in corso. Nel mondo sono migliaia i protocolli in fase di studio e solo l'AIFA fino ad oggi ne ha approvati ben Chiediamo quindi che si faccia, nel più breve tempo possibile, una sintesi di questi protocolli e si definisca un unico protocollo e linee guida unitarie per i nostri medici del territorio. Ad oggi le persone morte di Covid in Italia sono 112.374; di queste faceva parte Annamaria, la mia amica e maestra di vita. Molte di queste probabilmente potevano essere salvate, se avessimo utilizzato dei protocolli di presa in carico domiciliari più definiti. In medicina la prevenzione resta sempre l'arma più potente e più importante. Nel caso del Covid la prevenzione è certamente rappresentata dalla profilassi vaccinale. Noi davvero speriamo che aprile, come ha detto il commissario Figliuolo, sia il mese della svolta nella campagna vaccinale, ma prevenzione vuol dire anche prevenire le complicanze della malattia e mettere in atto una presa in carico precoce delle cure domiciliari. Siamo ancora in guerra e su questo campo di battaglia muoiono ancora troppe persone. Come in tutte le guerre però la chiave è risolvere prima il conflitto, perché la vittoria più grande è prevenire la guerra.

Ha fatto alzare una senatrice che è infortunata e ha il tutore. Non mi sembra né educato, né corretto. *(Applausi)*. CIAMPOLILLO *(Misto)*. Le ho chiesto se potevo. Mi ha detto di sì. Nell'ordine del giorno, presentato con il collega Martelli, relativo al potenziamento delle cure domiciliari Covid-19, al fine di prevenire e ridurre il carico sulle strutture ospedaliere, si è chiesto, tra l'altro, di valutare l'utilizzo di terapie alternative, come l'uso del CBD quale rimedio agli effetti letali del Covid-19. L'uso di tale principio attivo è già riconosciuto in Italia, essendo un farmaco prescrivibile e dispensabile dal Servizio sanitario nazionale, disponibile in farmacia. Tra le proprietà del CBD vi è anche quella di essere un potentissimo antinfiammatorio naturale, come attestato da numerosi studi scientifici citati nell'ordine del giorno. Già un anno fa ho invitato il ministro Speranza e alcuni ricercatori di settore ad approfondire il tema. raccolto la disponibilità di alcuni giovani medici e studiosi, avendo preso personalmente contatto con una nota azienda farmaceutica olandese, senza purtroppo ricevere dalle istituzioni italiane il giusto interesse. Orbene, è recentissima la notizia della pubblicazione scientifica del Medical college of Georgia presso l'Augusta university, negli Stati Uniti, che attesta come il CBD riduca la tempesta citochinica innescata dal sistema immunitario, potendo così evitare, o comunque fortemente attenuare, i danni più gravi al tessuto polmonare per effetto della ventilazione artificiale. Tutto questo ricordando che il CBD, già positivamente adottato nella terapia del dolore, contrariamente a tutti gli altri farmaci attualmente utilizzati non ha alcuna controindicazione o effetto collaterale dannoso, potendo dunque essere somministrato anche ai pazienti più deboli. Sembrerebbe quindi che l'inammissibilità dichiarata in seduta, relativamente alla seconda conclusione dell'ordine del giorno, sia dovuta alla volontà di evitare una votazione su un argomento forse troppo ostico da affrontare, piuttosto che a valide motivazioni comunque non esplicitate, considerando che gli impegni chiesti al Governo riguardavano proprio il potenziamento delle cure domiciliari, con l'ausilio di terapie migliorative, come il CBD per i soggetti affetti dal virus. *(Applausi)*.

nonostante il richiamo fatto, lei ha continuato nell'atteggiamento per cui l'avevo richiamata, e pertanto esprimo nei suoi confronti la censura da parte della Presidenza.

**Il Senato approva.**

Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la mozione a mia prima firma, oggi all'esame dell'Assemblea, sottoscritta da rappresentanti della maggioranza e da senatori di diversi Gruppi parlamentari, che ringrazio sentitamente, ha lo scopo di innovare la didattica della matematica e di introdurre il pensiero computazionale e algoritmico nelle scuole, per garantire un prospero futuro alle prossime generazioni. In Italia è attualmente attestato un grave ritardo nel campo della formazione matematica, tecnico-scientifica e informatica, che ostacola il pieno sviluppo della potenzialità delle persone e la crescita economica e sociale del Paese. La mozione in esame è stata depositata nel 2019, accompagnata da un convegno che si è svolto in Senato, alla presenza di Ministri e con la partecipazione di illustri esperti. In questi due anni non è diminuita l'urgenza di un'azione in tal senso. Nel 2019 riportavo il dato dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) della Commissione europea, di due anni fa, in cui l'Italia risultava al ventiquattresimo posto su 28 Stati membri. In particolare, nell'indicatore capitale umano, ossia chi ha competenze nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Italia si posizionava al ventiseiesimo posto tra i 28 Paesi. L'anno successivo, nell'indice DESI del 2020 si è registrato un ulteriore peggioramento: l'Italia è scesa al venticinquesimo posto su 28, perdendo una posizione nell'indicatore; in particolare, nel capitale umano l'Italia si posiziona al ventottesimo posto su 28, ossia all'ultimo posto, perdendo ben due posizioni. La mancanza conclamata di conoscenze digitali riguarda tanto gli adulti quanto i giovani. Tali lacune colpiscono tanto le imprese, che rischiano di non poter cogliere le opportunità offerte dal digitale, quanto la pubblica amministrazione, che rischia di veder vanificato ogni tentativo di transizione digitale per mancanza di professionisti con comprovate conoscenze scientifiche, matematiche, computazionali e informatiche. Anche a livello di esercizio della cittadinanza queste carenze mettono le persone a rischio di non poter far valere pienamente e consapevolmente i propri diritti, in quanto impossibilitati a comprendere il funzionamento delle nuove tecnologie in cui quotidianamente siamo immersi, quali ad esempio quelle che hanno a che fare con la protezione dei propri dati personali, la videosorveglianza di massa, il riconoscimento delle *fake news* e altre. Una fetta di cittadini non è più in grado di interagire con la pubblica amministrazione digitale. La consapevolezza dell'importanza di acquisire una formazione tecnico-scientifica specifica è cresciuta nel corso di quest'anno di pandemia, ma questo non basta sicuramente per misurare i risultati che ci consentano di risalire la china. Per programmare un piano di uscita da questo livello medio scarsissimo nelle competenze digitali, va rimossa la causa che alla base limita il numero di studenti iscritti alle lauree in Troppi bambini e soprattutto bambine vengono condizionati da un pregiudizio: non essere portati per la matematica, una disabilità irrimediabile che li rende inabili alla comprensione della matematica per tutta la vita.

si chiede al Governo di assumere alcuni impegni, in primo luogo di continuare ad investire nel Piano nazionale scuola digitale, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse e con l'introduzione di metodologie innovative più efficaci di apprendimento della matematica e del pensiero computazionale e algoritmico, specialmente nella scuola primaria, ossia nell'età in cui si insidia nelle bambine e nei bambini il pregiudizio di non essere nati per la matematica. Inoltre è necessario potenziare nei gradi successivi dell'istruzione percorsi di formazione innovativi e multidisciplinari, in cui il pensiero umanistico e quello scientifico scientifico si compenetrano e si rafforzano a vicenda. Un maggiore raccordo con la realtà e la necessità di misurarla consentirà agli studenti di orientarsi verso le discipline scientifiche e la matematica, intesa come disciplina che aiuta a comprendere molti aspetti della quotidianità e con un approccio multidisciplinare affina e sensibilizza alla percezione estetica e incoraggia i giovani ad affrontare la complessità e le sfide presenti e future del mercato del lavoro continua evoluzione. Si impegna altresì il Governo a connettere tale rinnovata strategia nazionale di formazione con i settori del lavoro, del *welfare* e dello sviluppo imprenditoriale, culturale e artistico del nostro Paese, in modo che questo innovativo approccio possa rappresentare un volano per la crescita complessiva e strutturare dell'Italia. Infine, si chiede di garantire una formazione professionale dei docenti, in sinergia con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione del personale Ringrazio il Governo e tutta l'Assemblea per l'attenzione nei confronti di un atto che ritengo fondamentale per il presente e il futuro del nostro Paese e dei nostri cittadini.

Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, una delle più importanti scuole di pensiero della storia dell'umanità prende il nome dal suo fondatore, Pitagora, matematico, scienziato, politico e taumaturgo che considerava l'errore una colpa della quale ci si poteva liberare solo attraverso il sapere, una delle leve più importanti. Vorrei citare, a questo proposito, le parole del senatore Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, goriziano di nascita, proferite in una *lectio magistralis*: «Avremo l'occasione di porre finalmente la domanda: a quale prezzo i cittadini sono pronti a sostenere un consistente ruolo intellettuale, tecnologico e culturale del nostro Paese all'interno dell'Europa e del mondo?». Socrate asseriva come soltanto chi ammette la propria ignoranza può mettersi alla ricerca della verità. La consapevolezza di non sapere dovrebbe costituire la più aspra contrapposizione a chi reputa di non avere alcun bisogno di imparare o a chi rimane chiuso nella propria *turris eburnea*, pensando che il mondo finisca dove finisce la sua sfera di interessi o di saperi. La pandemia ha messo in evidenza molte delle nostre lacune, scardinato innumerevoli certezze, portato alla luce la voragine tra ciò che è e ciò che invece dovrebbe essere, soprattutto in quella che generalmente viene definita una scienza esatta, ma anche, in senso pratico, quanto ancora dobbiamo lavorare per modernizzare il Paese per affrontare la didattica a distanza o lo *smart working.* La mozione che ci apprestiamo a votare ben evidenzia la necessità di confrontarci con l'impreparazione in campo digitale, che costituisce una delle massime sfide del Next generation EU per porre le basi del nostro futuro *tout court.* Dirà ancora l'illustre collega Rubbia: «Non andrebbe dimenticato quanto siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui gli strumenti necessari per dischiudere i segreti più disparati della natura arrivano alla portata della nostra tecnologia (...). Ma per costruire bisogna conoscere e prevedere. E da qui l'essenziale e universale legame (...) tra la conoscenza e l'invenzione Una rapida evoluzione della tecnologia è certamente la caratteristica più significativa degli anni a venire», conclude Rubbia. Negli anni Settanta del secolo scorso un artista triestino sloveno, Edward Zajec, formatosi negli Stati Uniti, aveva cominciato a riflettere seriamente sull'uso del computer nell'arte. Oggi viene considerato il pioniere della *computer art* nel mondo. Nella sua opera, infatti, arte e tecnologia interagiscono in perfetta sincronia. L'Europa non comprendeva appieno, aveva invece compreso molto bene l'America, che gli ha offerto nel 1980 una docenza nel dipartimento della Syracuse University di New York di cui Zajec alla fine è stato professore emerito, con strumenti digitali messi a disposizione da un colosso mondiale. All'inizio pochi avevano compreso quali e quante possibilità esistono, infatti a Trieste Zajec dovette avvalersi della collaborazione di un ingegnere informatico. In seguito, però, il dialogo tra il calcolo, il colore e il suono divenne linguaggio attraverso il quale Zajec ha evoluto la propria ricerca della verità qual è l'arte attraverso l'algoritmo generativo e interattivo. Per decenni, dunque, il nostro Paese non ha voluto né saputo cogliere *in toto* le sfide che invece nel mondo, dagli Stati Uniti all'India, trovavano spazio attraverso la consapevolezza che il digitale e quindi la formulazione matematica sarebbe divenuto la lingua globale per eccellenza, l'investimento per il futuro dell'umanità non solo nel campo scientifico o pratico, ma anche in quello artistico. La ricerca ha un unico comune denominatore, che è quello di porsi le domande e perseguire il fine che non può essere altro se non l'imperativo categorico del dovere che rappresenta - dirà Kant - la necessità di compiere un'azione per rispetto della legge morale. Questo è il senso del nostro voto: ripensare il rapporto con ciò che non abbiamo saputo prevedere, tra cui la pandemia, e gli strumenti che ci servono per non rimanere indietro.

drammatica già prima della pandemia. L'Italia è sempre stata fanalino di coda nella formazione in queste discipline e ciò comporta che solo una percentuale residuale di studenti scelga di specializzarsi in questi settori. settori. Oggi come oggi, la situazione si è aggravata notevolmente a causa della pandemia in corso. Sono stati fatti molti investimenti nelle strutture, nelle dotazioni strumentali delle singole scuole, nelle connessioni e nell'edilizia scolastica, ma le soluzioni trovate non risolvono purtroppo i problemi dei *gap* di apprendimento degli studenti.

L'investimento va fatto sulla qualità della classe docente e sulla formazione continua nelle tecnologie informatiche e digitali che devono supportare e non sostituire la didattica in presenza. L'investimento va fatto per consentire che ogni studente sia messo nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti per la sua fascia d'età, attraverso la riduzione del numero degli studenti per classe e un presidio didattico di sostegno pomeridiano permanente. Si tratta di interventi strutturali che incidono sulla spesa corrente. Gli osservatori internazionali hanno certificato che in Italia gli studenti del quinto anno di liceo hanno nelle discipline matematiche le competenze dei ragazzi di terza media. Questa è la situazione prepandemia e sta a significare che i ragazzi italiani avranno molte meno possibilità rispetto a quelli degli altri Paesi europei di essere impiegati nei settori strategici per lo sviluppo della nostra società.

Si è pensato a tenere aperte solo le scuole dell'infanzia e del primo ciclo fino alla prima media, ma tutte le scuole devono rimanere aperte. Ormai bisogna convivere con la situazione pandemica e fronteggiarla con misure sul trasporto pubblico, sui tracciamenti e sulla profilassi. Bisogna ricominciare a vivere

dell'istruzione pubblica, perché a una classe politica incompetente che pensa solo a servire le *lobby* per garantirsi l'autoconservazione serve un popolo ignorante e senza prospettive di mobilità sociale. La qualità della scuola pubblica indica lo stato di salute di un Paese democratico, della politica e delle Istituzioni. Penso che la qualità della nostra scuola sia l'indicatore più evidente del livello raggiunto da questa classe politica e dirigente.

di conseguire due lauree simultaneamente. A studenti costretti a colmare i prerequisiti mancanti per poter frequentare con profitto i percorsi di laurea

e atteso da 500.000 aspiranti docenti per l'accesso ai ruoli dell'insegnamento. Per poter insegnare con efficacia, bisogna intanto avere delle serie competenze disciplinari, perché non si può insegnare ciò che non si conosce. Quello che si conosce, invece, si può insegnare e si può adattare alle migliori strategie di insegnamento che si rendono necessarie

del Governo, colleghi, una riflessione come questa sull'insegnamento della matematica potrebbe sembrare un meccanismo che in qualche modo va a incidere esclusivamente sul cosa insegnare e come insegnare negli anni della scuola dell'obbligo. In realtà, dovremmo spostare l'attenzione su altri due parametri molto importanti, uno dei quali rappresenta il contesto serale abituale di ognuno di noi: ormai, quando accendiamo la televisione la sera, vogliamo sapere l'indice dei contagi a che punto sta, il numero dei guariti, il numero dei contagiati; vogliamo sapere quante persone ci hanno lasciato. E sulla base di questi numeri, facciamo delle proiezioni:

da dove vengono? Come sono stati ricavati? In base a quale principio questo numero si sposta e oscilla tra un margine e l'altro? La domanda su ciò che è dietro il numero numero rappresenta la sfida intellettuale più importante per tutti noi. Ma, a dire il vero, pochi di noi - io stessa non credo di potermi assolutamente annoverare tra i competenti in questo - sanno esattamente quei numeri da dove vengono. La cosa certa è che quei numeri determinano le scelte che si prendono.

il ragionamento scientifico dietro il numero si imponga alla maturità oggi dell'adulto e, in prospettiva, alla formazione dei più giovani. Claude Bernard, un nome molto noto a tutti coloro che in medicina si sono occupati del passaggio da una mentalità forse più empirica a un ragionamento scientifico più serio, sostanzialmente diceva che il ragionamento scientifico nasceva dall'osservazione, dall'ipotesi che si faceva su quell'osservazione, dall'esperimento che si creava per verificare quella ipotesi, dall'analisi dei risultati che si ottenevano da quell'esperimento e dal ragionamento su quei numeri. È evidente che il ragionamento sui numeri era possibile solo alla luce della correttezza del ragionamento scientifico che c'era dietro, a tal punto che - è una frase che risuona molto in medicina - se non puoi dirlo con i numeri, non lo dire. numeri, non lo dire. Il paziente sta meglio o peggio rispetto a che cosa: al parametro della febbre aumentata o diminuita? C'è il parametro del dolore: ma quanto soffre di più e quanto soffre di meno? il parametro di un indicatore che viene dalla tabella delle analisi che hai richiesto e che dice se i globuli rossi sono aumentati o sono diminuiti?

Non sono delle indagini cliniche, sono anche un esame molto attento fatto sul DNA del virus, cioè sequenze che vengono misurate in un modo o in un altro. Tutto il nostro ragionamento ha questo fondamento, lo diceva già Pitagora molti secoli fa. Insistere sulla formazione della matematica è insistere sulla formazione logica, sul rigore, sulla precisione, sulla correttezza dei dati che escono dal «mi sembra», dal «secondo me», dall'opinione e si agganciano a una oggettività che diventa confrontabile. Questa è la ricchezza che noi vogliamo trasmettere alle nuove generazioni attraverso un maggiore e migliore insegnamento della matematica; più formazione scientifica per decidere con maggiore libertà,

anch'io intervengo su questo argomento, che mi sta molto a cuore. Sia durante la trattazione delle linee guida del PNRR, sia in tutto il lavoro che ne è seguito e che ha portato a un voto la scorsa settimana, uno degli elementi che è emerso è stata la necessità che la scuola italiana si concentrasse sulla formazione di competenze in campo scientifico, proprio per diminuire il divario rispetto agli altri Paesi. È emerso in quella sede ed emerge tutte le volte che si parla con il mondo produttivo, ma anche con il mondo delle istituzioni: servono maggiori competenze in campo scientifico e in campo matematico. Ben venga allora questa mozione, che accende un faro su questo su questo problema. Effettivamente la risposta può arrivare già partendo dalla scuola primaria. Si parla di STEM, cioè di insegnare, di insegnare, attraverso dei laboratori, la possibilità di avere un pensiero che finisce con una costruzione, usando la parte tecnica e la parte logica e stimolando una capacità di pensiero diversa; questo è assolutamente importante. In alcune scuole - capita anche nella mia scuola primaria, che frequentai tantissimi anni fa - è sviluppato ed è esercitato con particolare interesse il gioco degli scacchi, come sport, da parte dell'associazione sportiva legata a questa scuola, proprio per attivare quei processi logici

Ci sono insegnanti di matematica che mi raccontano, anche in altre realtà, come gli insegnanti stessi cerchino di capire quali sono gli alunni più portati e di avviarli a facoltà come matematica e fisica, proprio perché queste facoltà

Ci sono per esempio dei campi interessanti che forse meriterebbero perlomeno delle sperimentazioni; parlo della programmazione neurolinguistica, alcuni definiscono pseudoscienza, ideata da Bandler e Grinder negli Stati Uniti degli anni '70. Si tratta di un metodo che migliora la comunicazione e che induce un maggiore sviluppo personale. Tutto quello che facilita

c'è una generale convinzione, da parte della maggior parte degli studenti e delle persone, di non essere portati per la matematica. La maggior parte delle volte questa è una convinzione fondata sul nulla. Il principio, però, è che, se noi crediamo una cosa e continuiamo a dircela,

rinforza l'autostima e la convinzione di poter fare di più. Questo sistema di pensiero e di educazione, secondo me, dovrebbe trovare nella scuola il luogo ideale, sin dalle primarie. Pensate, infatti, alla gioia dei bambini quando riescono a raggiungere un risultato: si sentono dei campioni. Questo modo positivo di pensare il primo passo, anche con questa sperimentazione e questo modo citato nella mozione. È un modo per far ripartire il Paese nel verso giusto, verso un progresso, che non è un vezzo, ma una necessità. Nel nostro Paese, infatti, servono più persone laureate in matematica, laureate in scienze, laureate in ingegneria: perché il mondo produttivo lo vuole, ma anche perché è un modo per pensare e

Signor Presidente, Antonio Gramsci scriveva: «Il vecchio mondo sta morendo. Quello nuovo tarda a comparire. E in questo chiaroscuro nascono i mostri». Ecco, noi ci siamo trovati di fronte a questa crisi sanitaria, che ha fatto emergere drammaticamente una condizione di emarginazione, di diritti individuali mortificati dalle logiche di mercato logiche di mercato e ci sta imponendo, quindi, una riflessione molto profonda. Sullo sfondo di questa crisi sanitaria, noi dobbiamo quotidianamente fare i conti con la crisi climatica. Entrambe ci impongono una profonda riflessione e, da più parti, è sentita l'esigenza di un nuovo umanesimo, di riportare al centro l'uomo. Come può accadere ciò? Ciò può accadere con la consapevolezza, attraverso una fase di transizione, non solo ecologica o eco-sistemica, come piace chiamarla a me, attraverso una transizione socio-culturale e bioantropologica. In questa epoca di grande progresso tecnologico, di furore tecnologico, dobbiamo preoccuparci di mantenerci saldi al controllo di questo progresso veloce e, dunque, di mantenere l'uomo al centro. Consapevolezza nel senso di procedere in questa transizione con consapevolezza; che significa procedere con conoscenza, capacità di osservazione, di speculazione, di pensiero critico. È, dunque, anche questa la finalità di questa mozione: promuovere quel campo di studi che permetta all'uomo di governare questo processo di veloce progresso tecnologico e di non ritrovarsi in subordinazione, non solo per via dell'incapacità di governare i processi tecnologici, ma anche per la perdita di sue capacità cognitive e umane che rischierebbero di porlo al servizio della macchina e non alla guida della macchina. Dunque, è il momento di ritrovare e rinsaldare l'alleanza e la collaborazione tra scienza e umanesimo. ripensare, dunque, in questa ottica lo spazio scuola e i percorsi didattici affinché questa alleanza e collaborazione

perché la scienza ha bisogno dei filosofi e degli storici dell'arte. Le due discipline si devono compenetrare,

dell'umanesimo, Albert Einstein scrisse una lettera a Robert Thornton, un giovane docente che doveva preparare il suo primo corso di fisica e cercava sostegno in Einstein per mettere più filosofia della scienza possibile in questo suo corso. Non a caso esiste la filosofia della scienza. Einstein scrisse: «Una conoscenza dello sfondo storico e filosofico fornisce proprio quella indipendenza dai pregiudizi della propria generazione dai quali la maggior parte degli scienziati sono afflitti. Questa indipendenza determinata dall'analisi filosofica è - a mio giudizio - il segno di distinzione tra un semplice artigiano o specialista e un autentico cercatore di verità». Dunque, Dunque, partendo da questa mozione, noi prendiamo per mano di nuovo l'umanesimo e insieme ci proiettiamo in un futuro in cui dovremo sempre avere ben chiaro il nostro obiettivo; formare individui e cercatori di verità.

Vorrei iniziare da questa frase: «La matematica è il futuro. Ragazzi, avvicinatevi a questa materia, provatala, non abbiate paura. Vedrete che vi ripagherà, anche economicamente». Sono le parole di Giovanni Sebastiani, un matematico e ricercatore. Queste parole mi sembrano più che mai adatte per evidenziare il ruolo sempre più preponderante della scienza nella vita di tutti noi, soprattutto a partire dai giovani. Oggi sappiamo che i dati - li ha ricordati prima la collega Mantovani - non sono per nulla incoraggianti da questo punto di vista. riferiti, in modo particolare, al nostro Paese sulle competenze matematiche, tecnico-scientifiche e digitali del capitale umano. Se da un lato l'Italia ha conseguito buoni risultati nello sviluppo del 5G in quanto sono state assegnate tutte le bande pioniere e sono stati lanciati i primi servizi commerciali, dall'altro vi sono rilevanti carenze proprio sotto il profilo del capitale umano. I numeri sono preoccupanti. Riguardano la percentuale molto più bassa rispetto alla media europea, soprattutto della popolazione nella fascia di età tra

La percentuale per le competenze digitali superiori e per il numero di specialisti e laureati nel settore della tecnologia, dell'informazione e della comunicazione è molto al di sotto della media europea. Quindi, purtroppo, l'Italia detiene un primato negativo e questo ha conseguenze a livello economico e sociale che potrebbero creare enormi problemi anche rispetto alla nostra perdita di competitività rispetto ad altri Paesi europei (penso alla Spagna, alla Francia, alla Germania). Il rischio principale per le imprese è quello di non saper cogliere importanti stimoli e opportunità offerte dal digitale, ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale, perdendo inevitabilmente competitività e produttività rispetto ad altre Si sta ormai cristallizzando un divario sempre più evidente tra le richieste di lavoro delle imprese, sempre più focalizzate su profili predominanti nel settore tecnico-scientifico e digitale, e la competenza professionale dei candidati in questi stessi settori. Tutto ciò non fa altro che aggravare una situazione per le imprese italiane certamente non facile. Peraltro, il ritardo in questo campo si scontra anche con l'esigenza di ridurre sensibilmente la difficoltà di dialogo tra i cittadini e la pubblica amministrazione, nonostante gli sforzi di quest'ultima per adeguare le piattaforme digitali. Insomma, in questo quadro la pandemia ha imposto un massiccio ricorso alle tecnologie digitali per dare continuità a livello globale alle attività scolastiche e ad alcune attività produttive, ma, nello stesso tempo, ha evidenziato i nervi scoperti e dunque le profonde carenze in questi ambiti così cruciali. Dopo un primo periodo di incertezza, queste carenze, se non saranno affrontate immediatamente, potrebbero comportare il definitivo distacco sotto il profilo della competitività globale dagli altri Paesi cosiddetti virtuosi, con conseguenze economiche e sociali disastrose. Come la pandemia ha dimostrato, c'è sempre più penuria e quindi più richiesta di persone che sappiano leggere e analizzare i *big data*, che siano in grado di applicare i modelli matematici alla realtà, ad esempio per fare previsioni. Ci sono aziende in Italia che non trovano personale specializzato e, con tutta probabilità, in futuro la medicina, ma anche la psicologia e le scienze sociali, avranno necessità dell'integrazione delle scienze dure, perché sarà sempre più importante analizzare i fenomeni quantitativamente, utilizzando il rigore dell'approccio matematico. In altre parole, si impone più che mai una seria riflessione da parte di tutti noi affinché si possa nel breve periodo invertire la rotta, proprio a partire, a mio avviso, dai giovani, che sono la risorsa su cui è indispensabile puntare, se vogliamo effettivamente far ripartire il Paese, come ci ricorda ogni giorno anche il presidente Draghi. Le discipline scientifiche e digitali sono gli strumenti che abbiamo avuto a disposizione durante questa emergenza sanitaria e proprio i giovani non potranno fare a meno di riscoprirne l'importanza, perché durante la pandemia ne abbiamo visto concretamente gli effetti. Allo stesso tempo, è necessario muoversi in fretta, anche per sfatare il mito che la matematica e le competenze digitali siano appannaggio di pochi e siano magari non adatte alle donne. Sempre per adoperare le parole di Sebastiani in una sua recente intervista, si parla di matematici soprattutto quando esce fuori il genio di turno, l'eccellenza, il giovane che magari ha studiato ad Oxford, che ha quattro lauree. Così però passa un messaggio parziale: sembra che la matematica sia un affare di pochi; invece tutti se ne possono appassionare e innamorare. Incentivare i giovani, dunque, per ridurre il divario presente, sia a livello universitario, sia a livello di istruzione secondaria, tra percorso scientifico e umanistico-sociale, adottando politiche attive di formazione a livello scolastico, anche per rispondere in maniera adeguata alle richieste provenienti dal mercato. Contestualmente e parallelamente occorre muoversi anche in un'altra direzione per abbandonare i pregiudizi che abbiamo ancora oggi proprio verso l'accesso delle donne ai settori di studio scientifici. Bisogna fornire una possibilità di scelta e al contempo dimostrare che non vi devono essere preclusioni di alcun tipo - culturali o materiali che siano - all'accesso a questi campi di ricerca. A causa dei nostri pregiudizi, una donna deve affrontare difficoltà infinitamente superiori a quelle degli uomini nel condurre ricerche estremamente impegnative. Quando riesce comunque a superare gli ostacoli e a padroneggiare la materia, allora sembra che debba possedere più coraggio, un genio diverso, uno straordinario Anche in questo, nel linguaggio, nella capacità di vedere, di cogliere, di leggere le cose, forse dovremmo avere uno sguardo diverso, paritario. diverso, paritario. D'altra parte, abbiamo esempi grandissimi nella scienza, e le donne stanno andando avanti con grande forza ed entusiasmo. Il nostro compito, dunque, è quello di trasmettere al meglio la necessità di investire su queste materie affinché anche le nostre figlie possano avvicinarsi in maniera diversa. In conclusione, Italia Viva e PSI votano convintamente a favore della mozione perché sosteniamo l'istruzione e siamo convinti della necessità di guardare al domani in maniera lungimirante, proprio a partire dai giovani. La ripresa economica dell'Italia passa inevitabilmente anche per una trasformazione digitale che si incardina su tecnologie e competenze che abbiamo il compito di sviluppare e valorizzare.

alla didattica a distanza. Tuttavia, rilevare che molti docenti fossero impreparati nell'attuazione di questa metodologia didattica comprova

Io suggerirei tre approcci risolutivi: uno che riguarda la formazione dei docenti, l'altro che riguarda la formazione degli alunni e quindi i *curricula*; il terzo che concerne il rapporto tra la struttura del pensiero matematico e la struttura dell'azione e della lingua. Qualcuno ha già parlato della correlazione tra lingua e matematica; la scuola italiana da questo punto di vista è assolutamente arretrata. Viene sempre posta una linea di demarcazione tra la formazione umanistica e la formazione matematica, ma basta pensare a quelle che vengono ritenute le lingue morte, il latino e il greco, per notare come la struttura sintattica chiaramente richieda una logica. Per quanto riguarda la formazione dei docenti, oggi sapete chi può accedere, ad esempio, all'insegnamento della matematica per la scuola secondaria di primo grado, cioè alle medie? Coloro i quali possiedono la laurea in matematica, ovviamente, fisica, scienze naturali, chimica, astronomia, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze agrarie tropicali e subtropicali, discipline nautiche e scienze ambientali.

leggendo un articolo del «Corriere della Sera» del 2009, dal titolo «Meritocrazia»; «la conseguenza della estrema diversificazione del percorso formativo del futuro insegnante, in assenza di una forte coesione curricolare,

cioè il trasmettere il proprio sapere con l'attività didattica e quindi indurre al saper fare. Nel realizzare ciò, però, non si può prescindere dall'evoluzione del pensiero del bambino.

per poi arrivare, dalla secondaria in poi, al pensiero ipotetico-deduttivo, che è probabilmente quello logico, quello che poi porta al pensiero scientifico.

Nella formazione occorre assolutamente tenere conto di quello che è il costruttivismo e della necessità di portare l'alunno a costruire i propri saperi.

costruirlo, cioè renderlo tale sempre attraverso la costruzione da parte dell'alunno. L'alunno, secondo il costruttivismo, non apprende la realtà oggettiva. La realtà diventa oggettiva nella misura in cui egli la costruisce dentro di sé. Detto questo, per quanto riguarda invece il rapporto tra la lingua e la matematica, in conclusione, fare un esempio molto semplice. Nella risoluzione di un problema, se l'alunno non ha la capacità e quindi una conoscenza di base adeguata per l'interpretazione del testo,

Molte delle cause di cattiva riuscita in ambito scolastico sono legate a quelli che noi chiamiamo disturbi, ma che in realtà sono stili di apprendimento diversi.

come è molto chiaro in questa fase interessante di Governo - anche ascoltando gli interventi di oggi, che i nostri punti di vista rispetto a questo tema sono tuttora diversi e sono rimaste diverse le priorità. però provato a comporre un punto di vista, partendo anche da alcuni dati, che pure sono sempre discutibili e interpretabili. Ad esempio, diffido dal nostro sguardo verso il resto del mondo, come se là ci fosse tutto il bene e da noi ci fosse tutto il male: credo non sia così e ho la fortuna di partecipare ad un'assemblea parlamentare con 47 Paesi, dove ognuno assume esattamente lo stesso punto di vista, rivolto al proprio

modello e di modalità dell'insegnamento di questa materia fondamentale. Credo che dal dibattito di oggi alcuni di questi temi siano emersi in maniera molto forte. Visto che quella odierna è una giornata di citazioni, nello nello spiegare il perché del nostro voto favorevole a questo testo, vorrei partire anch'io da una citazione. Di solito non leggo mai, ma questa la vorrei leggere: «La matematica è stata «La matematica è stata il mio apprendistato alla rivoluzione, perché mi ha insegnato a diffidare delle verità assolute e delle autorità indiscutibili. Democrazia e matematica, da un punto di vista politico, si somigliano: come tutti i processi creativi non sopportano di non cambiare». È la citazione di un bellissimo libretto di Chiara Valerio, «La matematica è politica», che suggerisco a tutti di leggere, che rappresenta bene il mio e il nostro punto di vista rispetto alla mozione di oggi. Infatti la matematica è tutt'altro che l'insegnamento della certezza; certezza; è l'insegnamento dell'incertezza come una delle basi del mondo e della necessità di comprendere l'incertezza, di vivere nell'incertezza, di capire il senso della probabilità e di capire i meccanismi dell'interpretazione dei dati.

dinamiche distorsive possiamo apprendere. Com'è stato detto anche dalla collega Montevecchi, è anche fondamentale il tema di riuscire a dominare la *téchne,* invece che farcene dominare. È questa una grande preoccupazione dei migliori filosofi del Novecento europeo, che avevano percepito in tempi non sospetti (penso al filone ermeneutico, ad Heidegger e Gadamer) che la *téchne* avrebbe prevalso e schiacciato l'uomo. Oggi siamo dentro a quel tipo di paradigma e dobbiamo scegliere se vogliamo restituire alle generazioni future gli strumenti cognitivi, di conoscenza, per comprendere ciò che accade addosso a loro, attorno a loro, dentro di loro, oppure se rinunciamo a questa battaglia, per quello che succede all'interno di questi strumenti

ad esempio per ragioni economiche; una percezione che non considera i meccanismi degli algoritmi che le stanno dietro e si ferma alla superficie pensa che quello che sta vedendo è qualcosa di spontaneo, quindi

che vuole ad esempio tenere agganciate le persone, far prevalere alcuni contenuti rispetto ad altri, produrre risultati numerici (in particolare guadagni per alcuni), ma con elementi distorsivi e distruttivi della struttura della società. Un altro elemento che mi sembra emergere in maniera molto chiara da questo dibattito e che dobbiamo affermare in quest'Aula, dandogli anche il valore che ha, è che non esiste il contrasto tra umanesimo e matematica e noi, e noi, nel mondo, siamo quelli che possono affermarlo più di chiunque altro. Si usa tanto la parola «rinascimento». Cos'è stato il Rinascimento? È stato esattamente l'incrocio di questi due fondamentali saperi dell'uomo. Potremmo citare tante figure, ma credo ci basti probabilmente la più grande o una delle più grandi della nostra storia, Leonardo da Vinci, per capire cos'è il punto di equilibrio tra matematica e umanesimo. uno dei più grandi pittori, architetti, scultori, poeti e filosofi della storia dell'umanità, ma sicuramente un grande matematico, un grande scienziato e un grande studioso dell'armonia dei numeri nella natura,

in quella meravigliosa opera, di cui abbiamo discusso in 7a Commissione anche per la sua tutela, che rappresenta l'uomo del Rinascimento, in cui si ritrovano le proporzioni auree.

della transizione ecologica e del recupero di quest'armonia che, appunto, troviamo scritta nel grande libro della natura, come diceva Leonardo. Tutte queste questioni ci fanno dire che probabilmente tutti quelli di noi - e mi ci ritrovo - ai quali a un certo punto il verso di Antonello Venditti «la matematica non sarà mai il mio mestiere» ha suonato come proprio hanno incontrato insegnanti che non hanno saputo raccontar quello che ho cercato di riassumere in queste poche parole, cioè il fascino, la fantasia, la passione e la poesia contenuti in quel meraviglioso linguaggio che riesce a scrivere l'infinito

sul passato, ma diciamo - dati alla mano e sapendoli interpretare, perché è quello di cui stiamo parlando - che dobbiamo fare di più e meglio e dobbiamo lavorare anche sulla formazione *in *in itinere*, ad esempio, degli insegnanti. Questa è una fissazione del mio Gruppo politico, perché siamo convinti che i bravi insegnanti

perché la loro capacità di far apprendere passa dalla loro capacità di apprendere. Tutti sappiamo che i migliori insegnanti che abbiamo avuto - ce ne sono tantissimi nella scuola italiana - sono quelli che per loro scelta - molto spesso, bisogna per loro libera e volontaria scelta - hanno continuato a cercare stimoli, innovazioni e modi nuovi di insegnare. Vogliamo sempre di più che il nostro sistema dell'istruzione accompagni e dia gli strumenti anche economici a questi professionisti fondamentali per la tenuta e per lo sviluppo del nostro Paese, per continuare ad aggiornare le loro capacità durante tutto il corso della loro vita professionale. Tutti questi sono gli obiettivi - e sono tanti

affermiamo che è ora di chiudere questo tempo in cui il grande Paese della cultura, dell'arte, dell'Umanesimo e del Risorgimento possa essere pensato come quello in cui, per questa ragione, la matematica è una materia minore.

di grandi cambiamenti dal punto di vista delle strategie industriali, delle conoscenze e dell'innovazione digitale. Questa pandemia ha fatto sì che anche il nostro Paese, con tutti i ritardi che

ai colleghi - della separazione tra le discipline, con un approccio che non è mai stato interdisciplinare.

delle facoltà di fisica e matematica in tutti i nostri atenei (decapitazione che abbiamo poi dovuto recuperare con una certa fatica).

Perché credo che ancor di più dobbiamo fare in modo che la scuola formi i cittadini e dia gli strumenti e le conoscenze non solo affrontare il mondo di oggi ed entrare nel mondo del lavoro (che è assolutamente fondamentale), ma anche per avere gli elementi necessari ad essere cittadini pieni e poter scegliere in una società complessa come questa. Torno alla questione del momento di passaggio e di transizione tanto complicato. Rispetto alle grandi sfide che abbiamo davanti, che per quanto mi riguarda sono quelle di cambiare profondamente il modello di sviluppo (altrimenti la storia della civiltà umana avrà qualche difficoltà a sopravvivere), oggi ancor di più dobbiamo fare in modo

mi sono appuntato alcune parole: regola, metodo, razionalità, calcolo, oggettività, perseveranza e logica; perfino una parola che forse le riassume tutte: realismo.

elementi di più facile fruizione per tutti: l'improvvisazione, la semplificazione, il pregiudizio, l'emotività e la superficialità. Credo che uno dei mali della nostra epoca sia proprio questo: non riuscire a vedere la realtà per quello che è; non avere gli strumenti per analizzare i dati e comprendere le situazioni; di conseguenza, non essere nelle condizioni di risolvere i problemi. Lo abbiamo visto - è bene dircelo - anche in molte dichiarazioni di questa tragica fase pandemica espresse da parte della classe dirigente e di personalità evidentemente a disagio con il calcolo, refrattarie refrattarie al concetto di aumento esponenziale e in difficoltà di fronte alla necessità di fare equazioni coniugando dati. Tutto questo ha dei costi, che in questa fase tragica che stiamo attraversando si contano contano in termini di vite umane. La competenza matematica e quelle digitali sono necessità di quest'epoca, ma non solo: le competenze digitali sono figlie e frutto di quest'epoca. Lo si diceva prima, ed è verissimo: la tecnica non è mai neutra e in ogni epoca ha plasmato la mente della singola persona e, di conseguenza, le dinamiche sociali. Mai però prima di oggi una rivoluzione tecnologica come quella digitale, in così poco tempo e su una scala così vasta (il fenomeno è globale), ha ottenuto e determinato cambiamenti così profondi, sia nei singoli cittadini sia nelle singole società. È per questo che governare la rivoluzione digitale è il presupposto per dare un futuro al nostro Paese. E, per governare la transizione digitale e l'epoca in cui viviamo, non bastano la competenza tecnologica e l'educazione digitale, digitale, perché i numeri sono importanti, ma non sono tutto, sono necessari, ma non sono sufficienti, e vanno accompagnati alla cultura umanistica. I dati, per essere interpretati, non bisogna solo conoscerli e saperli leggere, ma anche saperli inserire in una logica ampia e globale. I *test* INVALSI citati nella mozione di cui discutiamo oggi, che gravemente mostrano carenze in termini di cultura matematica dei nostri giovani studenti, si accompagnano ad altri *test* INVALSI che non sono citati, perché non era questo l'oggetto della mozione, ma che denunciano un'altrettanto grave carenza dei nostri studenti in termini di conoscenza della propria lingua (l'italiano) e della storia. Non conoscere la storia, non per fare della facile retorica, vuol dire non conoscere sé stessi, quindi non essere nelle condizioni di affrontare il presente e di costruire il futuro, né di colmare

epoca). È evidente che il potenziamento dello studio della matematica deve accompagnarsi al potenziamento e all'integrazione dello studio della filosofia e della storia. il sapere scientifico da quello umanistico. Non è mai stato così; per millenni la cultura è stata una, un'unica cultura da Aristotele a Leonardo, fino a Goethe; è stata una e, all'interno di quell'unica cultura, quella scientifica ha contemperato la cultura umanistica ed entrambi gli emisferi di quest'unico globo del sapere hanno reso forte e libero l'uomo, perché senza cultura non si ha visione e percezione della realtà e, senza la visione e la percezione della realtà, non si costruisce nulla, ma si sopravvive e ci si lascia

(lo dico da semplice lettore). Mi pare che quella rivista abbia come obiettivo quello di alimentare il ritorno all'unicità del sapere, cosa obiettivamente meritoria. Mi ha colpito, nella sua banalità, un'affermazione in un recente editoriale della rivista in questione, cui si censura il fatto che molti intellettuali e molti uomini eruditi, di evidente e ampia cultura umanistica, siano soliti dire - e io mi metto tra questi, come figlio di una cultura umanistica, non certo come grande intellettuale - di non capire nulla di matematica. È un'affermazione che denuncia un problema; è una grande negligenza trincerarsi dietro un'affermazione di questo genere, superficiale e crea e rafforza il problema di cui ho parlato prima, perché, senza le qualità enunciate all'inizio del mio intervento (senza la regola, il metodo, la razionalità, il calcolo, l'oggettività, la perseveranza e la logica), la capacità di penetrare il mondo è ridotta; senza queste qualità,

Signor Presidente, colleghi senatori, ho dieci minuti di tempo, ma forse ne impiegherò meno per motivare il voto convintamente favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alla mozione in discussione, che intende impegnare il Governo a potenziare in diversi ambiti l'insegnamento e la conoscenza matematico-scientifica. Colleghi, questo potenziamento è necessario e indispensabile per i nostri giovani, per le nostre imprese e per i nostri cittadini, per essere preparati e competitivi, nonché cittadini attivi in una società in cui l'approccio tecnico, scientifico e digitale è - e

Quello che forse non abbiamo detto abbastanza e che ritengo, invece, si debba dire è che abbiamo una grande responsabilità: quella di non interrompere il processo di evoluzione, culturale e scientifica alla base del quale, dall'origine dei tempi, sta la matematica.

che, non a caso, derivava da *máthema*, scienza, che a sua volta deriva dal verbo *manthánein*, imparare. Da qui i *mathematikói*, vale a dire gli inclini a conoscere. Fu lui, Pitagora, a scoprire le relazioni matematiche che sono alla base della musica, dell'arte e delle proporzioni che dettarono - e dettano tuttora - la creazione di grandi opere architettoniche come i templi greci o gli spettacolari affreschi della Cappella Sistina di Michelangelo, che tutto il mondo ci invidia. Quest'ultimo è un affresco che deve la sua bellezza alla perfezione matematica con cui fu studiato e realizzato. Uno studio dettagliato avrebbe infatti dimostrato che il vero segreto della portentosa armonia tra le parti, che rende così bilanciati ed equilibrati gli affreschi della Cappella Sistina, è in realtà l'uso sistematico e voluto della cosiddetta sezione aurea. Possiamo definire quest'ultima come quel miracolo di proporzioni fra le parti parti insito nella natura stessa, che gli studi matematici hanno permesso di scoprire e quindi di applicare alle creazioni dell'uomo, con risultati di una magnificenza unica. Che dire, poi, di Leonardo e del suo genio? Dai suoi scritti, dalle sue sperimentazioni, dalle sue opere e dai suoi dipinti è evidente quanto abbia nutrito per i numeri e il calcolo un particolare interesse, ritenendo che dietro di essi vi fosse la possibilità di creare strade nuove, ancora sconosciute, sconosciute, in grado di portare la conoscenza dell'uomo verso una più ampia profondità. Ritornando a Pitagora, non dimentichiamo la scoperta della scala musicale, anch'essa basata su proporzioni matematiche e, a sua volta, base delle composizioni dei musicisti di ogni tempo. I legami tra il linguaggio musicale e i princìpi matematici sono indissolubili. Per questo, nella storia dell'uomo, la matematica e la musica le troviamo spesso unite indissolubilmente. Non solo: nell'anno di Dante non possiamo non ricordare quanto l'opera che lo ha reso celebre sia legata ai numeri e alle leggi matematiche nelle sue proporzioni. Le tre cantiche, formate da trentatré canti con strofe di tre versi, le cosiddette terzine, sono solo un esempio di come la matematica abbia condotto e ordinato la sua opera letteraria. Si potrebbero fare tanti altri esempi, a dimostrazione di quanto la matematica sia legata a ogni aspetto della vita, dell'arte, della quotidianità e delle nostre attività, anche sportive, in cui le regole e i campi da gioco, siano essi grandi o piccoli, sono realizzati e studiati in base a precise proporzioni e leggi matematiche. Ieri sera, cari colleghi, sono andata a riguardarmi quel bellissimo e attuale cortometraggio che la Disney ideò nel 1959, in cui il simpatico personaggio di Paperino fa un viaggio attraverso il mondo della "matemagica", in cui entra con il fucile, ma che, grazie allo spirito di avventura che lo accompagna, scopre quanto sia meraviglioso e sorprendente. Conclude il suo viaggio cercando di aprire con curiosità una serie di porte, quelle del sapere e delle possibilità che può offrire il futuro. Felice, Paperino, conclude che solo la matematica ha le chiavi per aprirle. Perdonatemi questa visione romantica della matematica, ma sono fermamente convinta che dobbiamo smettere di dire e dirci di non essere portati per la matematica, scusando con questa frase la nostra pigrizia nell'applicarci a una materia che, come abbiamo visto, è indispensabile e alla base di ogni nostro sapere, di ogni oggetto che usiamo nella quotidianità di ogni spazio, come quello di quest'Aula, studiata e organizzata secondo precise proporzioni geometriche e matematiche. Per questi motivi, abbiamo la responsabilità di continuare a coltivare e valorizzare il sapere matematico e scientifico che dall'inizio dell'umanità sta alla base di tutto e ci è stato tramandato dagli studiosi e dagli artisti di ogni tempo e che non può essere slegato dagli altri saperi. Possono essere diverse da quelle di una volta le metodologie con cui si applica la matematica. Oggi il nostro strumento è digitale e diventa sempre più indispensabile prenderne coscienza e acquisire le conoscenze necessarie per il suo corretto utilizzo. engineering and mathematic* (STEM), ovvero scienze, tecnologie, ingegneria e matematica, ancora meglio i licei STEAM, che aggiungono anche l'arte, per formare i nostri giovani. Ben vengano adeguate formazioni, ancora meglio se obbligatorie, per i docenti.

in un istituto paritario. Ne sono molto fiera e spero veramente che qualche componente del Ministero dell'istruzione possa essere presente.

gentili senatrici e senatori e onorevole rappresentante del Governo, ringrazio innanzitutto la senatrice Mantovani, che da anni si occupa dei contenuti riportati nell'atto oggi in discussione, e tutti i firmatari della mozione, utile a favorire l'innovazione della didattica della matematica, del pensiero computazionale e algoritmico e delle competenze digitali nelle scuole. Lo Skills outlook scoreboard dell'OCSE mostra, purtroppo, che la popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale sia nella società sia sul posto di lavoro.

Le aziende europee registrano difficoltà nel reclutare personale esperto in tali ambiti per una grave carenza di queste figure. L'Italia è in grande ritardo. Per quanto riguarda le persone in possesso di una laurea in informatica, il nostro Paese si posiziona ben al di sotto della media dell'Unione europea, con solo l'uno per cento sul totale dei laureati, contro il 3,5 dell'Unione europea. C'è anche un'importante differenza con l'Europa per quanto riguarda il ruolo delle donne: nel 2020 solo l'1,2 per cento delle lavoratrici si è specializzato in informatica, contro l'1,6 della media europea;

per quanto riguarda gli insegnanti, quelli italiani - non certo per colpa loro, ma per una mancanza di programmazione efficace - risultano meno preparati rispetto ai colleghi europei e utilizzano le nuove tecnologie molto meno di altri lavoratori con istruzione terziaria. Tutto ciò ha origine nelle lacune dell'attuale insegnamento della matematica nelle nostre scuole, tema spesso sottovalutato negli scorsi anni e che questa mozione ha il merito di mettere al centro del dibattito politico e istituzionale. Il punto da cui partire è l'importanza dell'alfabetizzazione matematica, ossia della capacità di un individuo di ragionare matematicamente e di formulare e utilizzare il ragionamento e il linguaggio della matematica per risolvere problemi di una varietà di contesti del mondo reale. Citando infatti la professoressa Lorella Carimali, autrice del libro «L'equazione della libertà», la matematica è lo strumento per intuire, immaginare, progettare, dedurre, controllare, verificare, misurare e quantificare fatti e fenomeni della realtà. Aiuta le persone a conoscere il ruolo che tale disciplina gioca nel mondo e a formulare giudizi e decisioni ben fondati, necessari ai nuovi cittadini del XXI secolo. Svilupperò brevemente ancora tre concetti: la matematica è creatività, la matematica è per tutti, la matematica è libertà. La matematica è creatività, è questione di immaginazione e di curiosità, quella che porta a vedere oltre la visione comune delle cose. I matematici sono curiosi e creativi. La creatività matematica è la stessa dell'artista dinanzi alla tela bianca. Infatti, i matematici hanno immaginato i buchi neri molto prima che gli astronomi ne trovassero traccia. Anche il bosone di Higgs è stato teorizzato matematicamente nel 1964 e la sua dimostrazione fisica è avvenuta nel 2012, negli esperimenti Atlas e CMS condotti con l'acceleratore LHC. Nel 2013 Peter Higgs e François Englert sono stati insigniti del premio Nobel per la fisica per la scoperta, che in realtà era del 1964, quarantanove anni prima: era semplicemente una scoperta matematica. La matematica è per tutte e per tutti noi. Essa, però, è legata ad un pregiudizio molto forte, che sia per pochi eletti e che per capirla occorre essere dotati di un *quid* dalla nascita. Non è in realtà vero: non esistono persone negate in matematica; esiste solo un pregiudizio che viene continuamente tramandato nelle scuole e, a volte, nelle famiglie. Questo è un danno mostruoso che facciamo alle nostre bambine e ai nostri bambini. La matematica - come ho detto - è creatività e rappresenta uno stimolo per migliorare la nostra capacità di imparare. Abbiamo quindi bisogno di queste attitudini nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, per riprenderci dal baratro in cui siamo caduti. Un quarto degli italiani abbandona lo studio della matematica e la percentuale degli analfabeti funzionali è la più alta d'Europa. Pertanto, si deve lavorare affinché la matematica venga percepita come per tutti e non solo per un'*élite*, rimuovendo i pregiudizi che tutt'oggi si instillano nelle nostre bambine e nei nostri bambini. Con questo nuovo approccio la competenza matematica può diventare una competenza di cittadinanza, fondamentale per la realizzazione personale e professionale dell'individuo. La matematica è infine libertà, che allarga lo sguardo all'infinito e all'universo. I matematici sono in grado di trasferire il rigore del loro ragionamento scientifico nella vita di tutti i giorni. Un vero matematico è sempre pronto a verificare ogni fatto e ogni informazione, è libero dagli istinti, è capace di superare pregiudizi e tabù. Colleghe e colleghi, la mozione in esame contiene alla base tutti gli elementi che ho citato. Prevede lo stanziamento, nell'ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, di adeguate risorse e l'introduzione di metodologie innovative più efficaci di insegnamento e apprendimento di tali materie e successivamente delle delle discipline STEAM e dell'educazione digitale. Prevede, inoltre, il potenziamento di percorsi di formazione innovativi a tutti i livelli, per l'orientamento degli studenti verso le discipline scientifiche, incluso il pensiero computazionale, algoritmico e la matematica. Tra gli impegni mi pare importante sottolineare quello che prevede di connettere tali rinnovata strategia nazionale di formazione con i settori del lavoro, del *welfare* e dello sviluppo imprenditoriale, culturale e artistico del nostro Paese, in modo che questo innovativo approccio possa rappresentare un volano per la crescita complessiva e strutturale dell'Italia. In conclusione, senatrici e senatori, voglio citare il filosofo e matematico Bertrand Russell, che sosteneva come la matematica, vista nella giusta luce, possiede non soltanto verità ma anche suprema bellezza: una bellezza austera, come quella della scultura.

che potrebbe diventare il più importante volano per la ripartenza del Paese e anche la leva essenziale per realizzare il miglior modello di rigenerazione urbana, configurandosi peraltro come strumento sostanziale della transizione ecologica, aiutando nel contempo a far ripartire l'economia e il lavoro in maniera virtuosa. Per evitare che una iniziativa così speciale possa poi, nella pratica, rivelarsi al di sotto delle aspettative e ci si possa ritrovare a non utilizzare *in toto* gli investimenti assegnati anche all'interno del Piano nazionale di ripresa semplificarne l'applicazione, come mi sembra sia volontà unanime del Parlamento. Signor Ministro, il mercato delle costruzioni vale 180 miliardi di euro, tre quarti dei quali generati da recupero edilizio.

Per questo oggi le chiediamo di valutare l'eventualità di consentire al maggior numero di utenti possibile l'opportunità di accedere al *bonus*, superando alcuni passaggi burocratici, come quello della doppia conformità di quegli edifici che presentano difformità interne veniali - quindi non nella sagoma esterna e né in situazioni gravi - tra i titoli edilizi di oggi e quelli risalenti alla costruzione, che alla fine sono solo figli della storia; considerando valide le asseverazioni che riportino gli estremi del titolo edilizio e la data di esecuzione dell'opera; ampliando i margini di tolleranza per regolarizzare le difformità o non prevedendone la dichiarazione, per la quale è già sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori in regime di edilizia libera, per non fermare la possibilità di intervenire su condominio. Grazie usando un intero capitolo di spesa previsto nel PNRR, riterremmo opportuno chiederle di valutare l'estensione del superbonus agli immobili considerati strumentali all'attività di impresa, alberghi, agriturismi, baite e rifugi di montagna. In ultima istanza, signor Ministro, sempre in ottemperanza alle linee del PNRR, le chiediamo che il Governo valuti la possibilità di procedere alla semplificazione a regime di tutti gli interventi edilizi di efficientamento energetico sotto un'unica aliquota del 75 per cento, prevedendo la durata della detrazione in cinque anni, oltre al cosiddetto sconto in fattura e la cessione del credito. La ringrazio tanto dell'attenzione e della disponibilità.

mediante un accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 36 del testo unico, oppure mediante il ripristino della situazione legittima con demolizione o altre misure; altrimenti si deve fare una procedura di fiscalizzazione dell'abuso

mi impegno a parlare al più presto con i Ministeri coinvolti e a darvi la risposta più opportuna possibile. Per quanto riguarda il secondo quesito sull'estensione del superbonus, mi impegno altresì ad avviare una riflessione col Ministero dell'economia e delle finanze, che in questo caso è più direttamente interessato. Sottolineo - giusto per completezza visto che abbiamo cominciato a rifletterci ieri che la misura in questione è stata introdotta con lo scopo principale di favorire interventi di riqualificazione profonda sotto il profilo energetico e sismico degli edifici residenziali, che rappresentano un ambito su cui concentrare gli sforzi anche nel Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, la *long term strategy* e la *renovation wave*. L'ampliamento della platea dei beneficiari anche agli edifici strumentali di imprese potrebbe risultare più complessa da conciliare con l'obiettivo di concentrare risorse pubbliche dove possono produrre maggiori risultati. Lavoreremo su questo. Adesso mi impegno ad aprire questa discussione con il MEF e vi saprò dire in tempi più rapidi possibili. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di procedere alla riforma delle detrazioni fiscali connesse agli interventi edilizi, in considerazione della strategicità del comparto costruzioni,

Fino a tali date il superbonus potrebbe operare insieme alle consuete detrazioni fiscali dedicate al settore (*bonus* casa, ecobonus, sismabonus, *bonus* facciate), ad oggi tuttavia limitate al 31 dicembre 2021. Per il periodo successivo potrebbe essere considerata una revisione coordinata del sistema delle detrazioni fiscali ad oggi esistente, con un approccio integrato che consentirebbe di ottimizzare tempi e costi degli interventi. La revisione del quadro normativo potrebbe tenere conto dei vincoli di bilancio e prevedere congiuntamente tutti questi profili, valutando, ad esempio, diverse aliquote di detrazione in funzione delle *performance* generali raggiunte da ciascun edificio. Concludo dicendo che il sistema delle detrazioni edilizie potrebbe, inoltre, continuare ad essere affiancato da strumenti di provata efficacia, come quelli della cessione del credito e dello sconto in fattura con procedure adeguate anche per le piccole e settore. In conclusione, mi impegno ad aprire subito questa discussione e vi farò sapere al più presto. Signor Ministro, la ringraziamo molto per la sua apertura, per la sua disponibilità e per la condivisione delle tematiche rispetto a temi che ormai sono diventati di sensibilità generale. Lei oggi guida un Ministero, quello della transizione ecologica, davvero strategico per contribuire a realizzare una visione generale del Paese che coniughi il rispetto dell'ambiente con il benessere complessivo dei cittadini (sociale, personale ed economico). Oggi risparmiare energia e realizzare gli efficientamenti a spron battuto sarà determinante per la ripresa del Paese, per adempiere alle direttive europee e perché finalmente, come dicevo, la sensibilità è cambiata. È tuttavia necessario che il Governo e il Parlamento tutto, che ne coadiuva l'azione, siano al fianco dei cittadini e delle imprese,

premesso che per noi naturalmente l'emergenza sanitaria è prioritaria

per programmare già le riaperture con un calendario preciso per i ristoranti, per le scuole, per i cinema, per i teatri e comunicassimo già oggi agli interessati quali sono le date di riferimento per la ripartenza, credo che faremmo un buon servizio per chi oggi vive una condizione economica di grande difficoltà e sicuramente saremmo nelle condizioni di farlo senza rischiare nuove ondate, proprio grazie a una campagna di vaccinazione che crediamo sarà efficace nelle prossime settimane.

quindi, parlerò a braccio e magari dirò qualcosa di non esattamente politicamente corretto. Ritengo che, in merito a questa esigenza assolutamente condivisa, dobbiamo appoggiarci - come lei ha richiamato nell'apertura del suo intervento - al principio della sicurezza. Questo principio della sicurezza sanitaria è in via di evoluzione anche grazie al dispiegamento della campagna vaccinale. Purtroppo, come è evidente a tutti, i progetti originari non sono stati puntualmente rispettati. Non siamo qui per discutere sulle responsabilità, anche rimesse - per e agli *stop and go* relativamente ad alcuni vaccini attualmente in uso. Il requisito di una ragionevole proiezione temporale del dispiegamento della politica vaccinale è il prerequisito per dare certezze; altrimenti il rischio è di dare, al contrario, incertezze. Abbiamo già sperimentato questo in occasione della riapertura degli impianti sciistici. Certamente tutti i colleghi senatori ricorderanno quel caso in cui poi la retromarcia ha costretto in qualche modo gli operatori a sopportare danni addirittura ulteriori e superiori rispetto a quelli derivanti da una mancata apertura. La volontà da parte del Governo, già in questi giorni, è di prendere effettivamente sul serio quell'impegno scritto nel decreto-legge circa la possibilità di avere delle riaperture anticipate nell'eventualità epidemiologici, certificati ovviamente dal comitato tecnico-scientifico, lo permettessero. Stiamo quindi facendo questo tipo di valutazione,

e l'intenzione di dare certezze e non di creare ulteriori incertezze, come magari avvenuto nel recente passato.

Signora Presidente, mentre accade quello che prima abbiamo sentito e il Paese deve fronteggiare la pandemia, purtroppo con risultati inferiori a quelli di altri Paesi europei, accade anche che quasi un milione di persone ha perso il posto di lavoro, certificato dall'Istat, e che il 45 per cento delle imprese italiane è a rischio, e molte a rischio di acquisizione straniera. In questo quadro si inserisce una questione importante, che riguarda proprio il settore su cui era rinata l'industria italiana, cioè il settore delle automobili, che ancora oggi, con l'intera filiera, produce milioni di posti di lavoro, se guardiamo a tutto l'indotto e alla filiera degli stabilimenti. Ebbene, è accaduto che nel frattempo si è realizzata quella che era stata annunciata come una fusione paritetica tra FCA, cioè la gloriosa FIAT italiana con la Chrysler, e il gruppo francese della Peugeot. Si parlava di fusione paritetica e invece scopriamo, dopo la fusione, che non è fusione, perché è una vendita alla Peugeot, e non è paritetica, perché la *governance* è a maggioranza francese, compreso l'amministratore delegato, indicato dai francesi, e compresi i sindacati, due presenti nel consiglio amministrazione, uno espressione dei sindacati francesi e l'altro espressione dei sindacati statunitensi. Nel frattempo, sappiamo che il *management* nominato dal nuovo amministratore delegato della Stellantis è a maggioranza francese. Nel frattempo, stamattina, dai giornali che nello stabilimento di Melfi si progetta la chiusura di una linea di produzione: si comincia a chiudere gli stabilimenti italiani. Ebbene, a fronte di questo sappiamo anche che la stessa *holding* ha messo in vendita il gruppo Iveco ai cinesi

una fusione o una vendita? Una *governance* paritetica o meno? Era stato comunicato che lo Stato francese, dopo la fusione, avrebbe aumentato le quote? Secondo: perché il Governo non mette in campo Cassa depositi e prestiti per acquistare una quota pari a quella che detiene lo Stato francese, garantendo che anche gli stabilimenti e la filiera italiani siano protetti da eventuali ristrutturazioni? Terzo: il Governo cosa intende fare con Iveco,

condivido il fatto che la politica industriale, con riferimento al settore dell'*automotive*, necessiti di una generale e profonda rimeditazione, che passa per il supporto non solo alla domanda, ma anche all'offerta, strumento indispensabile per garantire una seria politica industriale e incentivare gli investimenti nel Paese. miliardi e miliardi di euro per via nazionale e anche attraverso il *recovery plan* per promuovere la mobilità sostenibile di autobus e veicoli commerciali, poi si fa fatica a non immaginare un'offerta produttiva industriale italiana che tenda a soddisfare questo tipo di domanda; altrimenti andremo a comprare inevitabilmente all'estero, magari in Cina. Proprio un adeguato supporto al sistema industriale rappresenta la premessa per evitare operazioni di delocalizzazione o acquisizione di imprese nazionali, che altrimenti in molti casi, come quelli citati dagli interroganti, si vanno a configurare quali operazioni di natura privatistica, che rientrano nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia negoziale delle imprese coinvolte e che non rientrano nell'ambito delle fattispecie per le quali è possibile l'esercizio dei poteri speciali, soprattutto quando si tratta di operazioni intracomunitarie. Così è stato per le operazioni che hanno dato luogo all'attuale assetto del gruppo Stellantis. Dapprima si è infatti verificata la fusione tra FIAT Chrysler Automobiles e Peugeot. Il 25 settembre 2020 il gruppo di coordinamento istituito dalla normativa sui poteri speciali ha ritenuto la citata operazione vigente non oggetto di obbligo di notifica. La successiva cessione ad Assist Digital SpA da parte di FCA Italy SpA di una quota pari al 51 per cento del capitale sociale di FCA Customer Service, società attiva principalmente della fornitura di servizi di *customer care*, è stata oggetto di analisi e in sede di Consiglio dei ministri si è deliberato il non esercizio dei poteri speciali, con delibera del 18 dicembre 2020, per assenza dei relativi presupposti. Veniamo però al futuro. Per quello che attiene al gruppo Iveco, così come per Comau S.p.A. e Teksid S.p.A., citate dagli interroganti, allo stato attuale non risultano notificate operazioni che potrebbero dar luogo all'esercizio dei poteri speciali. Se e quando le operazioni aventi ad oggetto le predette società venissero intraprese, saranno prontamente avviate le iniziative istruttorie da parte del gruppo di coordinamento per valutare la possibilità di esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, anche alla luce del recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179 del 18 dicembre 2020, che individua ulteriori beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Come sa sicuramente il senatore Urso, all'interno di Iveco operano tanti settori di attività e di produzione, alcuni anche in qualche modo connessi all'industria della difesa.

ceduto ai cinesi, cioè l'ipotesi di opporre il *golden power*, non solo perché riguarda anche una materia della Difesa, ma anche perché l'intreccio tra parte civile e militare è tale che, ove fosse scorporata la parte relativa alla Difesa, la parte civile comunque non sopravvivrebbe. Ringrazio il Ministro anche per le informazioni che ci ha dato sul gruppo FCA e sulla fusione. Mi permetta di dissentire perché con la norma di legge, che peraltro abbiamo introdotto nel cosiddetto decreto liquidità, è prevista anche la possibilità di intervenire laddove si tratti di soggetti dell'Unione europea. Tale norma di legge è stata prorogata al 31 giugno grazie ad un nostro emendamento approvato in quest'Aula. Quindi, forse, qualcosa in più si poteva fare

Aggiungo inoltre che è un problema di politica industriale. Ne conveniamo con lei e con lei vorremmo finalmente delineare una politica industriale che non riguardi solo questo settore. Pensiamo alla siderurgia, pensiamo all'industria del bianco e ai gruppi che stanno chiudendo come Embraco

di uno Stato stratega che sappia indirizzare la politica industriale del suo Paese, sia laddove deve resistere, come nel settore delle auto, delle acciaierie, nel bianco e negli elettrodomestici, sia laddove può attuare una politica attiva, e pensiamo alla rete (cioè al digitale) o all'energia verde. Di questo Stato stratega noi vogliamo far parte, perché apparteniamo insieme al nostro amato Paese, cioè al sistema Italia.

addetti su produzioni alternative che dovrebbero essere avviate da aprile 2022. La chiusura degli impianti *cracking* del petrolchimico di Marghera, secondo le organizzazioni sindacali, avrebbe pesanti ricadute sulle produzioni a valle del sito, causando un drammatico effetto domino di chiusura e dismissioni, con grave pregiudizio per il futuro di un comparto strategico per l'economia locale e nazionale. Ricordo che gli stabilimenti di Ravenna, Mantova e Ferrara, che con Porto Marghera formano il quadrilatero della chimica, risulterebbero direttamente coinvolti dalla chiusura del suddetto impianto,

milioni necessari per il potenziamento delle banchine portuali per l'approdo di navi criogeniche atte a rifornire i siti di Ferrari e Ravenna. Ciò avverrà, però, dopo la chiusura. L'ENI finora non ha motivato le proprie scelte e non ha reso noto il proprio piano industriale per i prossimi anni, dal quale comprendere le prospettive future del sito di Porto Marghera e dei siti produttivi di Ferrara, Mantova e Ravenna in termini produttivi e occupazionali.

Relativamente ai siti di Ravenna, Mantova e Ferrara non si hanno notizie di progetti specifici di rilancio o di riconversione della produzione. La vicenda, per la sua rilevanza complessiva, necessita della rapida costituzione di un tavolo nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico con il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente interessati e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia Lombardia e Veneto. Signor Ministro, siamo qui a interrogarla per sapere quali siano le valutazioni del Ministro sui fatti riportati e se intenda adoperarsi per istituire il tavolo nazionale presso il Ministero finalizzato ad affrontare e risolvere rapidamente la vicenda descritta, per salvaguardare la continuità operativa dei siti produttivi di Porto Marghera, Mantova, quali iniziative intenda assumere per garantire che siano realizzati i progetti più volte annunciati dall'ENI, ma mai realizzati. Inoltre, quale sia il piano industriale di ENI anche relativamente ai siti di Mantova, Ravenna e Ferrara, che deve essere mantenuto e non solo annunciato e come l'ENI intenda relazionarsi con gli *stakeholder* discutendo con trasparenza le proprie politiche industriali.

Alla luce della paventata chiusura da parte di ENI del *cracking* di Porto Marghera, del timore di ricadute in tutto il quadrilatero della chimica, che include Ferrara, Mantova e Ravenna, il Ministero dello sviluppo economico sta monitorando la situazione per approfondire le strategie industriali che si vorranno perseguire nell'ottica di salvaguardare il settore e garantire la piena trasparenza. In tale contesto, la società coinvolta ha comunicato di aver impostato un piano che guarda al futuro e che vedrà la realizzazione di iniziative industriali basate su tecnologie innovative volte a una sempre maggiore sostenibilità, strutturate con la massima attenzione per l'occupazione e le competenze presenti sul territorio. In particolare, ha assicurato che sta proseguendo il confronto con le parti sociali e istituzionali e che Porto Marghera è considerato uno dei siti fondamentali della propria strategia di transizione energetica che la porterà al completo abbattimento delle emissioni generate da processi industriali e prodotti finali al 2050. Con il progetto di trasformazione di Porto Marghera, la società ha comunicato che verranno tagliate oltre 600.000 tonnellate annue di emissioni di CO2. La stessa ha ricordato che il percorso verso la decarbonizzazione ha avuto inizio nel 2014, proprio con la messa in produzione della bioraffineria di Venezia, la prima al mondo nata dalla conversione di una raffineria tradizionale che, insieme a quella di Gela, ha visto aumentare nel 2020 le lavorazioni complessive del 130 per cento. È un cammino nel quale ENI investire complessivamente nel prossimo quadriennio circa 4 miliardi di euro nei processi di trasformazione. La società ha segnalato che il piano finora delineato punta ad aumentare la capacità della bioraffineria, grazie al nuovo impianto per la produzione di idrogeno da gas metano che si aggiungerà agli investimenti già in corso, finalizzati a renderla totalmente *palm oil free* entro il 2023 e a realizzare nuovi impianti di chimica - settore strategico per ENI - in un'ottica di specializzazione per lo sviluppo dell'economia circolare. In particolare, il progetto prevede la realizzazione entro il 2024 di un nuovo impianto Versalis per la produzione di alcool isopropilico, le cui principali applicazioni sono nella farmaceutica e nella produzione di disinfettanti e cosmesi. In un'area dell'ex petrolchimico, l'ENI, con la sua società ambientale, realizzerà un impianto che produrrà bioolio, destinato al settore navale o utilizzato come biocarburante di termoliquefazione nella frazione organica dei rifiuti solidi urbani. inoltre allo studio la creazione del primo polo dedicato al riciclo meccanico avanzato delle plastiche, il cui sviluppo è uno dei pilastri della strategia di Versalis. Porto Marghera rappresenta pertanto un sito di elezione nell'ottica di fornire al mercato prodotti sempre più sostenibili e di alta qualità. L'evoluzione del sito implicherà la fermata degli impianti di *cracking* e aromatici di Versalis a partire dalla primavera 2022. In questa fase, prima della fermata, Versalis garantirà l'operatività degli impianti di sicurezza, nel rispetto delle norme, nonché la conferma di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di *asset integrity* e di ispezione e collaudo previsti nei prossimi mesi. L'*hub* logistico Versalis rimarrà uno snodo centrale per la fornitura di materie prime per le realtà industriali di Ferrara e Mantova, alle quali il rifornimento sarà garantito con continuità. Sono già in corso elementi di consolidamento per aumentare la flessibilità e l'affidabilità. Approfittando della presenza qui del collega ministro Cingolani, concludo dicendo che chiaramente la materia in relazione al decreto-legge all'esame del Parlamento sarà peraltro trasferita nelle competenze del nuovo Ministero che si occupa di transizione ecologica. Il tavolo richiesto dai colleghi senatori che hanno presentato l'interrogazione sarà sicuramente incardinato e il Ministero dello sviluppo economico, naturalmente in collaborazione con quello della transizione ecologica ed energetica, darà il proprio contributo.

lì accanto a lei c'è anche il Ministro della transizione ecologica e i Ministri qui presenti sanno benissimo quanto il nostro Gruppo sia attento a questo tema. Riteniamo che, per esempio, anche su Porto Marghera e su tutti i siti collegati vada fatta transizione,

perché non basta l'enunciazione dei principi o immaginare date protratte nel tempo; bisogna capire quali e quanti soldi ci sono, su quali settori e con quali tempi, con quali ricadute occupazionali, per quale trasformazione dell'economia e con quali garanzie, perché la sostenibilità ambientale deve stare in piedi con quella economica e anche sociale. Vede, signor Ministro, non vorremmo per esempio che si continuasse a dire che a Porto Marghera si farà si farà per esempio *waste to hydrogen*, collegato al riciclo della plastica, ma solamente meccanico e non chimico, perché è del tutto evidente che, se questo manca, la trasformazione di Porto Marghera e dell'indotto in grandi *hub*

*(Misto)*. Signor Ministro, come sappiamo, l'Italia è in forte ritardo rispetto alla Francia nella realizzazione di un polo per la produzione di vaccini con investimenti sia pubblici che privati. La Francia si è mossa con largo anticipo, da circa cinque-sei mesi, ed è già in grado di avviare sin d'ora una sua produzione di vaccini. Nel corso di un recente vertice il Ministro ha dato mandato di individuare le ditte in grado di partecipare alla produzione di vaccini in conto terzi entro l'autunno 2021, spiegando di voler mantenere il massimo riserbo sulle aziende interessate. Fonti del Mise hanno certificato che già molte aziende dell'industria farmaceutica italiana sono pronte a partecipare alla fase di infialamento e finitura dei sieri, mentre solo alcune avrebbero le capacità per produrre anche il principio attivo. Il Governo è dunque al lavoro per verificare la possibilità dell'uso di bioreattori esistenti o di produrli *ex novo*, con l'intenzione di stanziare risorse e organizzare i siti, individuando come Regioni il Veneto, il Lazio e la Puglia, con tempi che variano da quattro Il Ministro ha affermato anche che sarebbero stati allocate importanti risorse a tale scopo, pari complessivamente a una cifra tra i 400 e i 500 milioni di euro, da inserire nel decreto-legge sostegni e in un prossimo nuovo decreto. Chiedo al Ministro se la prima *tranche* delle risorse del decreto sostegni, pari a 200 milioni di euro, sarà distribuita considerando la clausola del 34 per cento della spesa ordinaria prevista prevista dal cosiddetto decreto Mezzogiorno o, in subordine, se il Ministero terrà conto delle maggiori risorse da attribuire al Mezzogiorno attraverso i fondi UE, come previsto dagli indicatori del regolamento europeo del 12 febbraio 2021; se anche nel decreto che si appresta a firmare per la seconda *tranche* saranno rispettati gli stessi criteri; se non ritenga, infine, nell'ambito della realizzazione di un programma di sviluppo industriale, che gli stabilimenti per la produzione di vaccini vengano individuati in più Regioni del Mezzogiorno, atteso che in Puglia l'unica azienda, la Lachifarma, nel proprio stabilimento in Provincia di Lecce ha già investito 20 milioni di euro con risorse proprie, senza contributi. Quindi, pur rispettando la volontà del Ministero di mantenere il riserbo sulle aziende coinvolte, chiediamo in sostanza il criterio territoriale di allocazione delle risorse. PRESIDENTE.

una precisazione per quanto riguarda gli stanziamenti intervenuti su questa materia. In primo luogo, ricordo che con il recente decreto-legge sostegni, attualmente in corso di conversione, sono stati stanziati 200 milioni per la previsione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore biofarmaceutico italiano e per gli interventi complementari e funzionali (articolo 20, commi 7 e seguenti). Dette risorse sono funzionali all'incentivazione della produzione in Italia di vaccini destinati, sì, al superamento dell'attuale crisi epidemiologica, ma soprattutto alla prevenzione e al contrasto di futuri analoghi eventi. Le stesse si aggiungono a risorse già destinate da precedenti provvedimenti amministrativi alle medesime finalità. Risultavano infatti già stanziati 200 milioni di euro per il finanziamento di contratti di sviluppo aventi a oggetto programmi del settore biomedicale e della telemedicina, nonché tecnologie e servizi finalizzati alla prevenzione delle emergenze sanitarie. Tale dotazione è stata recentemente integrata, con decreto del 5 marzo 2021, attualmente in corso di perfezionamento, di ulteriori 150 milioni di euro. Con il medesimo decreto sono state peraltro definite nuove modalità di attuazione volte a rafforzare il sostegno prestato nell'ambito dello strumento. Sul punto tengo a precisare che le risorse sono quelle attualmente stanziate a legislazione vigente e che le stesse potranno essere successivamente incrementate in ragione dell'utilizzo dei fondi resi disponibili dall'Unione europea. Le nuove modalità di attuazione di cui al citato decreto del 5 marzo 2021 prevedono infatti la possibile applicazione allo strumento dei contratti di sviluppo delle disposizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (cosiddetto *temporary framework*). È stata disposta, per quanto di interesse, l'applicazione delle disposizioni specificatamente previste per lo sviluppo e la produzione di medicinali e prodotti direttamente connessi al Covid-19.

sostenere la realizzazione di investimenti "produttivi" in maniera più tangibile (75 per cento delle spese per le infrastrutture di prova e 80 per cento delle spese per gli investimenti produttivi), indipendentemente dall'ubicazione degli investimenti e dalla dimensione dell'impresa richiedente, superando, in tal senso, gli stringenti vincoli derivanti dall'ordinaria disciplina degli aiuti di Stato attualmente applicabile a tale categoria di investimenti; concedere le predette agevolazioni nella forma di sovvenzione diretta o anticipi rimborsabili. L'applicazione delle predette disposizioni è attualmente al vaglio della Commissione europea per la necessaria preventiva approvazione. Sul piano delle modalità di individuazione dei siti potenzialmente interessati, la priorità attualmente è il contrasto alla pandemia in corso e, pertanto, gli interventi che dovranno essere in una prima fase privilegiati sono quelli che consentono la più rapida operatività degli stabilimenti coinvolti, proprio al fine di garantire la produzione in Italia dei vaccini disponibili. In tale quadro, sono tutt'ora in corso le attività di verifica dei siti potenzialmente interessati, che dispongano delle idonee tecnologie e che siano disponibili alla immediata riconversione dei processi produttivi. L'individuazione di detti siti prescinde, pertanto, dalla relativa ubicazione territoriale, dovendosi fare riferimento piuttosto ai suindicati parametri e alla capacità produttiva, aspetti sulla cui base dovranno essere allocati gli incentivi e pertanto distribuite le risorse disponibili sulla base dello strumento dei contratti di sviluppo, previsto dalla citata norma primaria.

quello che abbiamo fatto al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Governo, è individuare quei siti produttivi che, nell'arco di un tempo ragionevolmente breve, dai quattro ai dieci mesi, fossero idonei ad attuare un processo di riconversione produttiva, indipendentemente dalla localizzazione. È un processo molto complicato, perché richiede la compatibilità delle tecnologie, dei brevetti e delle licenze che sono a disposizione delle aziende che sono sono diventate ormai note alle cronache quotidiane (Moderna, AstraZeneca, Pfizer, CureVac) con gli impianti esistenti. Quindi, in questa prima fase, l'urgenza è relativa agli impianti che sono potenzialmente in grado di riconvertirsi. Diverso è il discorso che comunque il Governo, nell'ambito delle risorse che saranno stanziate successivamente, intende attivare la creazione di quel polo polo vaccinale e della ricerca biomedica che sicuramente rispetterà le indicazioni e le percentuali che ha ricordato il senatore De Bonis nella sua interrogazione.

necessario per realizzare questi investimenti e probabilmente anche in aree già fertili da un punto di vista industriale, che possono già vantare un'esperienza nel campo farmaceutico. C'è un'eccezione in Puglia e c'è già chi è avanti e ha fatto degli investimenti. L'occasione di questa crisi pandemica

cercare di ridurre queste diseguaglianze che il Covid ha accentuato e confido che le azioni del Governo tengano in debito conto gli investimenti futuri per il Mezzogiorno.

È altrettanto oggettivo che il commissario Figliuolo ha dato un impulso diverso al piano vaccinale, come ricordava bene prima anche il senatore Faraone, ma nonostante queste premesse è evidente che l'immunità di gregge, tanto utile e tanto necessaria, è ancora lontana. Credo che l'autonomia vaccinale, per un Paese come il nostro, rappresenti una priorità e un aspetto fondamentale. Apprendiamo anche del buon esito del quarto tavolo che è stato tenuto al Mise per la produzione diretta o per conto terzi del vaccino. Questa è evidentemente una sfida fondamentale, per la ripresa economica e per l'intensificazione del piano vaccinale, attraverso la disponibilità dei vaccini. quale sia lo stato dei fatti in merito alla produzione italiana di vaccini anti-Covid-19 e quali tempi siano stimati per il raggiungimento di una vera e propria autosufficienza vaccinale, che veda l'Italia in un ruolo di rilevanza nella ricerca e nella produzione anche nell'ambito di eventuali scenari futuri. PRESIDENTE.

ciò che è stato fatto, in termini pragmatici, è capire quello che oggi esiste e che può essere convertito, come dicevo prima rispondendo alla precedente interrogazione, per far in qualche modo sposare

i brevetti, da parte dei noti *big* che ho richiamato in precedenza, siano resi disponibili, con forme di *partnership*, a questi produttori nazionali. A livello europeo, il commissario Breton ha avviato questo tipo di incontri tra i produttori italiani e i detentori di licenza.

indurle a valutare la possibilità di costituire in Italia dei poli produttivi, a beneficio dell'Europa e anche per i mercati non europei.

che l'Italia e l'Europa non debbano avere la capacità di rispondere alle sfide, a diversi pericoli, a diversi virus e a diverse varianti del Covid che oggi conosciamo, per non ritrovarci spiazzati, come ci siamo trovati in questa circostanza. il nostro Governo, a tutti i livelli, a partire dal Presidente del Consiglio, è fortemente impegnato in questa prospettiva che, lo ribadisco, non è tanto rivolta all'oggi o al domani, è rivolta magari al dopodomani. Dobbiamo però evitare che chi sarà su questi banchi e sui banchi del Parlamento tra due, tre, quattro o cinque anni, si ritrovi esattamente nella stessa situazione in cui ci siamo trovati oggi, ovvero nell'incapacità di rispondere alle attese, alle preoccupazioni e ai bisogni della nostra gente.

La valenza che questo può avere rispetto al suo progetto è evidente non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico, in termini produttivi e occupazionali. È evidente che questo tipo di atteggiamento avrebbe dovuto essere messo in campo molto prima, lo dico senza polemica: andava fatto molto tempo fa.

è sicuramente in una situazione complessa e per questo le siamo vicini. Il Ministro, però, deve garantire al massimo i livelli occupazionali. È il diretto responsabile dell'Alitalia attuale, quella che vola, quella in amministrazione straordinaria, ma fa parte nello stesso contesto di quel gruppo di Ministri che di concerto devono dare il benestare al piano industriale della nuova compagnia di bandiera. Le domande sono tante, ma cercherò di concentrarmi su poco e di essere anche chiara.

quasi spontanea: secondo me c'è un'altra proposta. I tecnici sanno che rinunciando a fette di mercato non si fa un piano di rilancio, ma sostanzialmente si rischia concretamente di volatilizzare la compagnia di bandiera. Questo Governo ha chiesto all'illustre commissaria Vestager, che parla tanto di concorrenza, di venire a indagare nel nostro Paese sul palese *dumping* all'interno del settore trasporto aereo? L'illustre commissaria Vestager, che parla tanto di concorrenza, ha mai indagato sugli aiuti di Stato attraverso incentivi e *co-marketing* falsi su tratte consolidate e non nuove? L'illustre commissaria Vestager si è mai chiesta come si possa pagare un biglietto 9 euro quando di tasse solamente se ne pagano 50? commissaria Vestager si ricorda il caso Tercas? Penso che noi ce lo dovremmo ricordare. Io penso solo che chi tratta con l'Unione europea dovrebbe avere in mente che noi dobbiamo avere un progetto Italia, un progetto Paese. La nostra compagnia, quella che sarà (la ITA

dipendenti più l'indotto, che a sua volta genera dipendenti nonché gettito? Questo è la compagnia di bandiera. La compagnia di bandiera porta organi, medicinali, radiofarmaci, porta aiuto e supporto alla Protezione civile. Vogliamo davvero spegnere completamente la speranza di avere un rilancio del settore del trasporto aereo? Io penso di no, signor Ministro, e confido nella sua posizione politica all'interno di questo gruppo di Ministri che di concerto devono dare il loro benestare a questo piano, auspicando che venga rifatto totalmente.

chiarezza a beneficio di tutti, perché forse non è molto chiara l'esatta ripartizione delle competenze. Il Ministero dello sviluppo economico risponde di quello che è rimasto, per così dire, della vecchia Alitalia con l'amministrazione straordinaria. Il progetto ITA è totalmente nelle facoltà e nelle prerogative del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha promosso la *newco* denominata ITA e che ha curato e sta curando naturalmente il piano industriale

Come è stato evidenziato dagli interroganti, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 79 della legge 17 marzo 2020, n. 18 e della conseguente costituzione alla società ITA per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo, sono state avviate ripetute interlocuzioni con la Commissione europea al fine di definire il perimetro della nuova società e l'acquisizione da parte degli *asset* di pertinenza di Alitalia attualmente in amministrazione straordinaria. Mi preme precisare che dette interlocuzioni non sono il frutto di una libera scelta, ma risultano imposte dalla legge nazionale che ha previsto la costituzione di ITA. Infatti, l'articolo 79, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2020, dopo aver previsto che per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci è autorizzata la costituzione della nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, prevede espressamente che l'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea. Inoltre, il comma 4 della richiamata norma dispone che il piano industriale presentato da ITA è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza e che la società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale tenendo conto della decisione della Commissione europea.

all'assenso da parte della Commissione europea. Non bastava tutto quello che già in qualche modo è previsto da parte delle normative europee, dalle direttive sulla concorrenza, ma il di cui anch'io facevo parte, anche se adesso sono al Governo, ha approvato una norma che impone al Governo di presentare il piano industriale e avere l'assenso della Commissione europea, altrimenti non può andare avanti. avanti. Lo dico perché le norme si approvano, si possono anche cambiare e questo naturalmente è rimesso alla vostra facoltà. In detto quadro, la Commissione non ha mai escluso la possibilità della costituzione di una compagnia di bandiera, ma il dialogo si è incentrato sull'analisi della regolamentazione di settore, della disciplina degli aiuti di Stato e dei requisiti, ivi compresa la cosiddetta necessaria "discontinuità", perché il nuovo soggetto non possa essere chiamato a rispondere della complessiva posizione debitoria della precedente compagnia. In particolare, i cosiddetti prestiti ponte, che sono stati in qualche modo illegittimi, credo che il 30 aprile dovrebbero in qualche modo essere restituiti o imputati a ITA. Nel contesto della trattativa, non sono emersi elementi per poter ravvisare un atteggiamento discriminatorio nei confronti dello Stato italiano. Anche la vicenda degli *slot* non appare al momento dissimile rispetto a quella in qualche modo imposta ad altri soggetti in ambito europeo

aerei limitato, il numero degli *slot* in qualche modo deve essere coerente. Questa è la posizione che ha la Commissione europea. Non va in ogni caso trascurato - questo è un altro elemento che tengo a sottolineare qui la complessiva operazione va valutata ed analizzata non solo nell'ottica della *newco*, ma anche nel pieno rispetto delle esigenze dell'amministrazione straordinaria di Alitalia, di cui è prevista l'acquisizione da parte degli *asset.* Qui ci sono dei creditori dell'amministrazione straordinaria. In base alle norme universali della *par In base alle norme universali della *par condicio*, i creditori in questo momento fanno ancora affidamento sull'amministrazione straordinaria (penso agli aeroporti, a chi rifornisce il carburante e ai dipendenti). In detto quadro è ferma intenzione del Governo adottare tutte le iniziative funzionali alla più celere conclusione delle trattative, che proseguono a oltranza anche in queste ore, anche in queste ore, nell'ottica di realizzare quanto prima un assetto che garantisca gli interessi dello Stato italiano, ma risulti nel contempo coerente con la disciplina europea, evitando possibili ricadute negative in termini giurisdizionali, che rischierebbero di minare l'operatività della compagnia proprio in fase di decollo. Nell'ambito delle trattative si stanno vagliando le più adeguate modalità realizzative della complessa operazione e anche, come ultima possibilità, quella di effettuare l'affitto di uno più rami d'azienda di Alitalia, nel rispetto del principio di discontinuità. Questa opzione

In ogni caso si vigilerà affinché le condizioni di operatività di ITA e delle correlate operazioni di acquisizione del patrimonio aziendale, anche tramite trasferimento da parte dell'attuale compagnia di bandiera, non siano meno favorevoli

lei ha parlato della crisi di Alitalia, che dura da anni. Ciò è noto; ci sono state tante campagne elettorali con Alitalia e vorrei evitare di farne un'altra. *(Applausi)*.

lo stabilimento Versalis di Brindisi, compreso nel polo petrolchimico situato nell'area di Pedagne e incluso nel perimetro del sito di interesse nazionale di Brindisi. Questo impianto è da sempre soggetto soggetto a un'attenzione particolare da parte dei cittadini e anche delle autorità locali, a causa di frequenti fiammate provenienti da alcune torce. Diciamo che l'impianto ha anche anche visto molti accenni sulla cronaca, per via di alcuni rilievi fatti dall'ARPA; c'è stato un periodo in cui il Comune di Brindisi ha deciso anche la sospensione dell'impianto di *cracking*. Adesso in che situazione siamo?

con l'azienda, al fine di implementare e rafforzare il monitoraggio necessario, che è stato già pattuito. Oltre a questo, un'altra cosa importante da fare per il territorio brindisino è che l'azienda deve garantire a stretto giro degli investimenti in *best available technology*, per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente. È inoltre necessaria una programmazione congiunta tra le diverse imprese del territorio, che coinvolga quindi non solo Versalis, ma anche tutte le altre industrie che operano nel brindisino, affinché ci sia la salvaguardia della resilienza del territorio e si garantisca un'adeguata transizione sia energetica che occupazionale ed ecologica. Signora Presidente, non è la prima volta che parlo di MPS, la più antica banca, inghiottita in un *crack* di 60 miliardi, tenuta ancora in vita dagli interventi degli azionisti e dello Stato, con infinite iniezioni di capitale, le cui condizioni finanziarie furono aggravate con la delibera n. 154 del 17 marzo 2008, firmata dal Governatore di Bankitalia, che autorizzava l'acquisto di Antonveneta con operazioni a debito fino a 9 miliardi di euro (il conto finale è stato poi di 17 miliardi), anche tramite strumenti ibridi e *bond* subordinati da appioppare al pubblico indistinto. sotto la guida di Mussari e nel 2012-2015 con Profumo e Viola, MPS ha illecitamente contabilizzato come investimenti in titoli di Stato 5 miliardi di euro di temerarie speculazioni in prodotti finanziari derivati, eseguite con Deutsche Bank e Nomura, con la finalità di occultare le perdite di altre operazioni di investimento (Santorini ed Alessandria). Ieri il tribunale di Milano ha reso note le motivazioni della sentenza di condanna per Profumo e Viola a sei anni di reclusione per le spiccate capacità a delinquere, pienamente consapevoli degli errori sui derivati e sul loro operato, il cui inganno sta nell'incetta di denari che si sarebbe da lì a poco perpetrata con gli aumenti di capitale, sussistendo pure un ingiusto profitto in favore di MPS, parsa navigare in migliori acque grazie al falso che ne ha accresciuto la percezione di affidabilità, non residuando dubbi e piena consapevolezza dell'erronea contabilizzazione a saldi aperti desumibile dal granitico compendio probatorio raccolto in plurimi e convergenti elementi di significativa pregnanza testuale. I giudici affermano che gli organi di vigilanza - Bankitalia e Consob - hanno assistito inerti agli accadimenti, limitandosi a insignificanti prese d'atto nella vorticosa spirale degli eventi, dalle allarmanti notizie di stampa fino alla *debacle* giudiziaria che un più accorto esercizio di controllo avrebbe certamente scongiurato. signora Presidente, ho presentato molte interrogazioni su MPS, tutte prive di risposta, col Governo azionista di maggioranza tramite il MEF, vero e proprio muro di gomma che, all'assemblea del 6 aprile, ha respinto l'azione di responsabilità promossa dal socio Giuseppe Bivona e dal fondo Bluebell verso Profumo e Viola e torna a chiedere le ragioni della mancata azione di rivalsa per i danni da 5 miliardi di euro verso le autorità vigilanti per omesso controllo e di tutti gli artefici dei 60 miliardi di buco nero

nella città di Barletta sono cominciati i lavori per la realizzazione di un supermercato accanto al fossato di un superbo castello angioino, su un'area tra le più sensibili della città compresa tra il castello, le antiche mura del centro storico e il mare; un'area a forte sedimentazione archeologica che esprime l'identità marinara della città; una cartografia cinquecentesca colloca proprio nei pressi del castello il molo di levante dell'antico porto dei canosini di epoca romana o addirittura preromana; un'area il cui pregio è stato riconosciuto dal decreto ministeriale 14 novembre 1974, dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il castello angioino in Comune di Barletta. La questione ha destato una diffusa contrarietà popolare. Il provvedimento autorizzativo appare regolare, ma proprio oggi sulla stampa leggo seri dubbi. generale vetusto lo ha consentito, laddove un piano urbanistico generale moderno avrebbe potuto impedirlo, anche attraverso perequazione. Poi manca l'attenzione verso il centro storico inteso come organismo vivo e complesso nel quale occorre tutelare le attività commerciali. Infine, la conservazione e la tutela di un monumento non possono prescindere dalla tutela del contesto socio culturale, storico, architettonico, ambientale e paesaggistico in cui esso è inserito. Lo afferma la Carta di Venezia del 1964. Mi appello al Ministero dei beni culturali affinché tuteli l'area in oggetto, i coni di visuale del castello e gli eventuali resti archeologici. Invito l'amministrazione comunale a rivalutare l'*iter* amministrativo; e considerare l'eventuale necessità di bonifiche ambientali nel sottosuolo, data la vicinanza di un'area dove insistevano depositi di carburante, e a vigilare sull'osservanza delle norme in tema di verde. Ultima *res*: auspico che l'amministrazione comunale e la proprietà si incontrino per una delocalizzazione perequativa che salvaguardi il diritto privato, ma soprattutto quello pubblico, della fruibilità socio-culturale, ambientale e paesaggistica dell'area. La bellezza ci salverà tutti.